dei voti che esprimeremo domani in Aula e devo chiedere a lei e al Presidente del Senato di effettuare un approfondimento, se necessario nella Giunta per il Regolamento, in maniera da evitare di inquinare la mattinata di domani con discorsi sulle procedure e di avere questa sera chiarezza di voto. Si tratta di un voto molto importante e penso sia interesse di tutti, Presidente, che siano chiarite procedure, termini e modalità nella giornata di oggi. Presidente, il senatore Calderoli ha presentato una proposta di risoluzione, che recita testualmente «Verificata la continuità della linea di politica estera

presentazione e nei termini di tale proposta di risoluzione. Presidente, penso sia doveroso che, nella circostanza, noi evitiamo che il Senato si impantani in procedure e modalità e che, rispetto al tema che abbiamo davanti, sia chiaro ai cittadini qual è invece la vera volontà del Senato. Mi consenta dunque di porre, con richiami

quale si verifica che la relazione che terrà il ministro D'Alema domani risponde a determinati requisiti. Presidente, non voglio dire, perché so di esagerare,

il senatore Calderoli avrebbe dovuto almeno aspettare che il dibattito iniziasse per presentare la sua proposta risoluzione; tuttavia, insisto fino ad un certo punto su queste obiezioni perché mi rendo conto

che sia data precedenza alla risoluzione accolta dal Governo. Solo in questi casi si pronuncia il Regolamento

e chiedo su questo una riflessione, se necessario anche della Giunta per il Regolamento. Un altro motivo mi fa sostenere questa tesi: sia per quanto riguarda l'emendabilità, sia in genere nella prassi parlamentare, per ogni strumento si comincia sempre a votare da quello più generale, perché ricomprende quello più particolare e lo assorbe.

Lei deve riconoscere che in Aula vi è stato un po' di trambusto quando, dopo il voto sull'ordine del giorno del senatore Calderoli su Vicenza,

essendo già avvenuta. Insomma, Presidente, occorre che siano messe a punto tutti questi aspetti, perché la votazione di domani non può essere affidata a giochi, giochini e trabocchetti. La questione è estremamente seria

che ho piena stima e piena fiducia del senatore Calderoli quando presiede la nostra Assemblea e aggiungo che il giudizio superlativo è poco, perché si rasenta la perfezione; ogni tanto, però, il senatore Calderoli (lo dico con simpatia) prende i panni dello zuzzurellone e introduce nella vita politica, con dichiarazioni o anche con risoluzioni, degli strumenti che creano qualche problema che è più vicino allo scherzo che non alla sede istituzionale nella quale ci

che, per evitare che, in una situazione così seria, si scada in una questione di giochi, giochini e trabocchetti, il Presidente del Senato debba applicare pienamente l'articolo 8 del Regolamento, quello che prescrive che il Presidente stabilisce l'ordine delle votazioni. Le chiedo di esercitare questo potere, in modo che dal voto escano, con chiarezza, per il Senato, per la Nazione e per la comunità internazionale, le linee di politica estera del Governo. Quindi, niente giochini, niente trabocchetti; mettiamo in condizione tutti di sapere effettivamente qual è la posizione della maggioranza, qual è la posizione dell'opposizione, qual è la posizione del Governo. Presidente, mi consenta di dire che, se si dà una risposta a tutte queste mie osservazioni, penso che facciamo veramente gli interessi delle istituzioni e dell'Italia.

l'intervento del collega Boccia, perché in qualche modo anticipa il dibattito di domani mattina. Per carità, lo fa con molto garbo legittimamente, ma mi pare di poter dire che anche giorni fa, quando c'è stato il dibattito sulla questione dell'ampliamento della base militare USA a Vicenza, il Presidente del Senato, con grande senso di responsabilità, ha messo ai voti le mozioni così come l'articolo 8 recita. Io non ho nulla in contrario la questione al Presidente del Senato, che ha senso di responsabilità e fino ad oggi lo ha esercitato, devo dire, in maniera del tutto condivisibile nel rispetto dell'articolo 8, ma il collega Boccia è andato oltre. Ora, qui siamo di fronte ad un dibattito politico molto serio, che fino ad oggi si è svolto al di fuori di quest'Aula, di quest'Aula, attraverso le televisioni di Stato e non, attraverso i giornali, attraverso manifestazioni di piazza (per carità, anche queste legittime), ci sono stati addirittura interventi di segretari di partito che hanno indicato al Ministro degli esteri, che domani deve venire qui in Senato a tenere una relazione, cosa dire e cosa non dire, quali argomenti usare e quali non usare.

La vostra maggioranza dovete cercare di tenerla insieme non attraverso le furbizie regolamentari (rispondo a lei con la stessa frase che lei ha rivolto a noi: senza furbizie), ma verificando se c'è una maggioranza

un modo assolutamente strumentale di aprire quest'oggi un dibattito che credevo iniziasse domani mattina. Se vogliamo che inizi oggi, il Gruppo di Alleanza Nazionale è totalmente disponibile a farlo.

pronunciata con garbo e con il sorriso sulle labbra, non può lasciare quest'Aula insensibile. Vede, collega Boccia, noi stiamo parlando di una risoluzione che questo Senato ha approvato

forse saremo di carattere allegro, ma la voglia di scherzare quando si vota e quando si discute degli impegni internazionali e di alleanze strategiche del Paese, non ci viene. Le ricordo una favola, quella del re nudo. Ecco, collega Boccia, forse quella risoluzione è servita a far vedere, sul piano politico, che il re è nudo. Le ricordo, collega Boccia, che lei ha parlato di tre posizioni che devono venire espresse in modo chiaro: quella del Governo, quella della maggioranza e quella dell'opposizione. Vede, Presidente, non sempre in quest'Aula giustamente le opinioni di maggioranza e Governo sono state equiparabili. In questo caso, siamo curiosi di sapere se le opinioni della maggioranza e le opinioni del Governo collimano, però rigetto con forza forza l'opinione dello scherzo, imputabile, tra l'altro, alla Presidenza attuale, e rimando al mittente, cioè alla maggioranza, la necessità di una politica chiara, che probabilmente non possiamo anticipare, ma non sappiamo se ascolteremo. Probabilmente, domani si parlerà di tutto, tranne che di Vicenza e questa sarà l'unica cosa che potrete fare per tenere uniti i pezzi della maggioranza. Detto questo, Presidente, credo che la Lega Nord si appronterà a un dibattito serio, senza alcuna voglia di scherzare, che parelatro ci è passata da quando questi colleghi hanno vinto le elezioni. finestra"). Senatore Boccia, credo che ci sia sufficiente prassi per darle risposte senza dover convocare la Giunta per il Regolamento, anche perché questi dotti dibattiti sul Regolamento e sull'ordine dei lavori spesso compaiono in occasione in occasione delle questioni pregiudiziali e allora bisogna approfondire meglio l'argomento. In ordine alla ricevibilità di risoluzioni, mozioni o ordini del giorno, al giudizio della Presidenza e il collega Calderoli può presentare, se sono ammissibili, qualunque tipo di risoluzione o mozione e poi rinviare al voto dell'Aula la valutazione del merito dello stesso. Sull'ordine del voto, lei giustamente ha citato specifici riferimenti a due fattispecie particolari previste dal nostro Regolamento, per cui si iniziano a votare quelle che hanno avuto il gradimento del Governo.

Infine, la ringrazio per le parole rivolte al Presidente: forse non conviene tenere il collega Calderoli in giro per l'Aula, ma conviene tenerlo alla Presidenza.

Oggi pomeriggio inizierà la discussione del decreto-legge sul recepimento di direttive comunitarie. Domani mattina, come già stabilito, avranno luogo le comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulle linee di politica estera

si svolgeranno con trasmissione diretta televisiva, a partire dalle ore 12,15. Nel pomeriggio di domani saranno discusse la proposta della Giunta delle elezioni in ordine alla costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzioni e due ratifiche di accordi internazionali, oltre all'eventuale prosieguo del decreto-legge sul recepimento di direttive comunitarie. Nella seduta antimeridiana di giovedì 22 febbraio sarà esaminato il disegno di legge recante modifiche al Codice di procedura civile in materia di procedimenti ingiuntivi. Nella seduta pomeridiana di martedì 27 febbraio avrà luogo la votazione, mediante schede a scrutinio segreto, per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro componenti supplenti della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti. Dopo la chiama iniziale, le urne resteranno aperte. Nella seduta antimeridiana di mercoledì 28 febbraio saranno discusse mozioni sulla politica ambientale. Sempre nel corso della prossima settimana saranno altresì trattati - ove conclusi nelle Commissioni competenti - il disegno di legge costituzionale, già approvato dalla Camera dei deputati, per l'abolizione della pena di morte e il decreto-legge per la prevenzione della violenza nelle competizioni calcistiche. Infine, i Capigruppo hanno convenuto che nella prossima Conferenza, da convocarsi nella giornata di martedì 27 febbraio, sarà stabilita la data di avvio dell'esame del disegno di legge recante modifica al Codice civile in materia di cognome del coniuge e dei figli.

recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani

il disegno di legge in esame reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 297 del 2006, recante disposizioni urgenti per il recepimento di direttive comunitarie.

In particolare, esso reca il recepimento delle direttive europee 2006/48 e 2006/49 del 14 giugno 2006, rispettivamente in materia di accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, nonché di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. Con queste direttive sono state recepite nell'ordinamento comunitario le raccomandazioni del cosiddetto Accordo di Basilea 2 in materia di regolamentazione prudenziale delle banche e delle imprese di investimento. Entrambe le direttive costituiscono la rifusione delle precedenti direttive quadro in materia, rispettivamente la direttiva 2000/12/CE e la direttiva 93/6/CEE. L'attuazione delle previsioni di tali direttive nell'ordinamento nazionale ha richiesto interventi a livello di norme di rango primario e secondario, da realizzarsi entro il termine di recepimento del 31 dicembre 2006. Sul piano legislativo, considerata la necessità e l'urgenza di rispettare tale termine, si è provveduto all'emanazione del decreto‑legge di cui discutiamo, con cui sono state apportate ai Testi unici bancario e della finanza le modifiche e le integrazioni necessarie ad adeguare la normativa interna di rango primario a quella comunitaria. La sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza, alla base dell'adozione del decreto-legge, è stata motivata con il fatto che il mancato recepimento tempestivo delle disposizioni delle direttive, che non costituiscono mera refusione e mera riscrittura delle norme preesistenti, avrebbe vulnerato gravemente il sistema Paese sia in termini di credibilità e immagine, sia sotto il profilo della *par* *condicio* di banche e di imprese di investimento italiane nei confronti dei loro competitori stranieri. Il provvedimento legislativo ha rappresentato il presupposto per l'adozione dei successivi atti di normazione secondaria, consistenti in una deliberazione del CICR da adottare su proposta della Banca d'Italia e nelle relative disposizioni di attuazione da parte della stessa Banca d'Italia. Affinché il termine del 31 dicembre 2006 risultasse rispettato, anche con riferimento agli atti di fonte *sub* primaria, già nelle more della formale emanazione del suddetto decreto legge, la Banca d'Italia ha trasmesso una proposta di delibera al CICR; per le ragioni di urgenza evidenziate, in luogo della delibera CICR, è stato adottato, con il ricorso alla procedura d'urgenza previsto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di Presidente del CICR. Il decreto è del 27 dicembre 2006 e reca il numero 933. Il decreto è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 22 gennaio 2007; in quella stessa *Gazzetta* *Ufficiale* ha trovato pubblicazione anche la circolare della Banca d'Italia n. 263 del 2006, che completa il complesso processo normativo di recepimento delle due direttive comunitarie all'interno del nostro ordinamento. Vorrei sottolineare brevemente la particolarità della catena normativa appena descritta; in cima a questa catena normativa c'è un accordo stipulato a Basilea tra le banche centrali e le autorità di vigilanza. Si tratta di un accordo che ha natura un po' originale; non è la prima volta che, in qualche modo, in base a quell'accordo - successe già con l'Accordo cosiddetto di Basilea 1 1 - viene redatta la direttiva dell'Unione Europea; la direttiva poi, in questa lunga catena normativa, viene recepita nell'ordinamento italiano con legge o con decreto legge di recepimento - nel nostro caso, con un decreto legge - cui seguono la delibera del CICR e la circolare a applicativa della Banca d'Italia.

accordo, del 2004 - è quella di pareggiare il terreno competitivo tra i diversi intermediari finanziari operanti nel mondo. In regime di libertà di movimento dei capitali c'è sempre il rischio che la differenza nella severità della disciplina a tutela della stabilità del sistema finanziario possa generare competizione al ribasso degli ordinamenti (competizione nel lassismo, dicono gli anglosassoni). Ciò vuol dire che la presenza di un diverso grado di stringenza delle regole in materia di stabilità finanziaria può determinare la localizzazione dell'attività di intermediazione nel Paese che Paese che utilizza le regole meno severe, più lassiste. Se questo avviene, i Paesi sono indotti a competere in lassismo, con regole sempre meno severe; il rischio complessivo è che si riduca il grado di stabilità del sistema finanziario mondiale nella sua interezza. Per evitare questa competizione al ribasso nella regolamentazione, ormai dal 1998, si prova a porre rimedio a questo con gli accordi tra le Autorità di vigilanza che poi, lungo la catena normativa che ho provato a descrivere,

che le banche dovevano rispettare in funzione dei rischi che si assumevano, secondo regole uniformi nel mondo che evitassero la competizione al ribasso. L'Accordo di Basilea 1 andava incontro a numerosi problemi, relativi in particolare al fatto che fatto che la classificazione del rischio era molto approssimativa e grossolana. Faccio un esempio: concedere credito ad un'impresa buona o ad un'impresa cattiva comportava la necessità dello stesso accantonamento di capitale, di capitale, ma in realtà, dal punto di vista economico, aveva senso imporre requisiti di capitale maggiori nel caso in cui il credito veniva concesso ad un'impresa meno buona. Quindi, uno dei primi criteri della riforma è quello di adeguare i requisiti patrimoniali in qualche modo all'effettiva rischiosità degli attivi bancari. Ciò comporta la necessità che le banche e gli intermediari siano in grado di classificare gli imprenditori di credito secondo il loro effettivo grado di rischio. Come sappiamo, se ne è a lungo discusso, sostanzialmente sono due gli strumenti utilizzabili a seguito

tipicamente le agenzie di *rating*, o il ricorso ai cosiddetti *rating* interni, cioè a modelli di valutazione del rischio interni alle singole banche che dovranno essere validati e in qualche modo convalidati anche delle Autorità di vigilanza dei singoli Paesi, quindi, nel nostro caso, dalla Banca d'Italia.

i soggetti di dimensione più rilevante, in particolare quei soggetti che affidano risparmi di grande dimensione alle banche, affinché preferiscano banche che siano maggiormente stabili. Si prevede dunque una disciplina delle informazioni che le banche devono rendere al mercato sulle proprie condizioni di stabilità in senso lato, che è poi l'obiettivo di un rafforzamento sistematico della collaborazione tra Autorità, necessario in relazione al fatto che la globalizzazione dei mercati finanziari procede molto velocemente. Quindi, anche la presenza di intermediari appartenenti a gruppi che operano in diversi Paesi del mondo rende necessario, ai fini di una maggiore efficacia nella vigilanza di stabilità, una forte collaborazione tra le Autorità di vigilanza. vigilanza. Quanto alla discussione che si è sviluppata in Italia sull'Accordo di Basilea 2, che comporta numerosi adempimenti da parte delle banche e rende a me pare più moderno il rapporto tra banche e prenditori di credito,

quanto riguarda gli adempimenti richiesti alle imprese, si fa più severa, in particolare, la trasparenza informativa richiesta alle imprese per venire incontro agli strumenti di valutazione del credito, di cui si doteranno le banche alle quali

prima delle riforme che ci apprestiamo ad introdurre nell'ordinamento italiano, concedere un prestito di 100 milioni di euro ad una singola impresa, ovvero concedere cento prestiti da un milione di euro a cento piccole imprese era indifferente, dal punto di vista dei requisito di capitale richiesti dalla disciplina di vigilanza prudenziale. Con le modifiche che saranno introdotte a seguito del recepimento dell'Accordo di Basilea 2, a parità di condizioni, sarà più conveniente fare cento piccoli prestiti, piuttosto che un solo grande prestito. È ovvio che ciò introduce, sotto questo particolare aspetto, un vantaggio e non uno svantaggio per le piccole imprese: noi sappiamo quanto le piccole imprese siano importanti e diffuse nel nostro Paese.

banca e della finanza, intervenendo solo dove è effettivamente necessario. Mi pare un'ottica ragionevole, tanto più che lo strumento del decreto-legge dovrebbe essere utilizzato proprio per introdurre modifiche strettamente necessarie al fine di fine di rispondere alle esigenze straordinarie di necessità ed urgenza dettate dalla Costituzione. Tuttavia - e su questo punto torneremo, perché ho preparato d'accordo con la Commissione un apposito ordine del giorno me pare che la quantità di interventi di modifica normativa introdotti nei testi unici della banca e della finanza, in particolare a seguito dell'attività intensa di recepimento delle modifiche normative introdotte nell'Unione Europea nell'ambito del Piano di azione sui servizi finanziari, sui servizi finanziari, ha fatto sì che i nostri Testi unici in materia bancaria e finanziaria presentino al proprio interno alcune incongruenze, alcune definizioni non sempre chiarissime in qualche caso alcune contraddizioni e comunque alcune complicazioni di difficile lettura. Credo sia necessario che complessivamente il Governo e il Parlamento mettano mano ad un riordino della disciplina nel settore del credito e della finanza, arrivando se possibile ad un Testo unico unitario del credito e della finanza, che realizzi un più stringente coordinamento tra le varie norme e se possibile una semplificazione delle stesse. Come dicevo, il decreto alla nostra attenzione non si occupa solo di aspetti finanziari, di modifica al Testo unico delle banche e della finanza: era contenuto nella versione originaria del decreto un articolo

questione. La norma è dunque diventata inutile e la Camera dei deputati ha fatto bene a sopprimerla. L'articolo 4 riguarda l'attivazione di poteri sostitutivi nei confronti della Regione Liguria. Si tratta della sospensione dell'applicazione di una legge regionale

per i giovani. È una norma necessaria: la costituzione dell'agenzia è la condizione per l'accesso a risorse comunitarie nel settore delle politiche giovanili e bisognava provvedere per tempo, in fretta, per evitare che alcune risorse finanziarie risultassero inutilizzabili per il nostro Paese. L'articolo 6 reca la copertura, che è relativa al solo articolo 5 di cui appena detto e che si riferisce alla costituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani, per i giovani, non essendo previsti oneri finanziari relativi agli articoli precedenti. In conclusione, a me pare necessario e utile che il Senato proceda all'approvazione del disegno di legge alla nostra attenzione. Forse, in astratto, alcuni piccoli aggiustamenti avrebbero potuto essere utili, ma l'urgenza di provvedere al recepimento delle direttive e in generale delle decisioni comunitarie

l'ottimo è nemico del buono e comunque, ripeto, ci troviamo di fronte ad un'attività di recepimento che presenta, soprattutto per la parte più consistente che riguarda l'adeguamento dei Testi unici bancario e della finanza, una qualità dei testi normativi più che buona e una regolamentazione che corrisponde

detto che l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, prevede che il Governo possa assumere provvedimenti con carattere d'urgenza necessari a fronte di atti normativi e a sentenze dell'Unione Europea, solo quando questi atti prevedano una scadenza che non potrebbe essere rispettata se si attendesse l'esame della Legge comunitaria dell'anno in corso.

intendo sottolineare che la decisione 1719/2006/CE, adottata il 15 novembre 2006, istituisce il programma «Gioventù in azione», che prevede una serie di interventi di lungo periodo, dal 2007 al 2013, per la formazione dei giovani, per cui non esisterebbe affatto il carattere di necessità e urgenza richiesto dall'articolo 77 della Costituzione, che giustificherebbe l'introduzione di questo articolo nel testo del decreto-legge in esame. sarebbe stato costituzionalmente più corretto, anche ai fini di una migliore valutazione degli interventi in questione, aspettare l'*iter* della prossima legge comunitaria. Con queste premesse, ribadita la non sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, nonché dall'articolo 78 del Regolamento del Senato, invito l'Aula, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, a non passare all'esame del decreto-legge n. 297 e ad esprimersi di conseguenza in sede di votazione. Signor Presidente,

soggiace, impiegato dal Governo per dare adempimento a una direttiva comunitaria, è stato ben regolato - come dicevo nell'illustrazione della pregiudiziale

politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità Europee e dell'Unione Europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso». Ebbene, gli articoli 1 e 2 del decreto‑legge in esame, che sostanzialmente - come ha appena illustrato il relatore - riguardano il recepimento di alcune normative in merito a Basilea 1 e Basilea 2, hanno in sé la motivazione e le caratteristiche di necessità e urgenza alla luce della succitata legge e, quindi, al riferimento costituzionale cui mi sono appellato.

in particolare, è stata cassata alla Camera dei deputati (pur rimanendo nel titolo del provvedimento) e riguardava l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti.

che le determinazioni della Comunità Europea abbiano uno spazio temporale iniziale nel 2007 e ultimativo nel 2013, indubbiamente non mi consente di pensare che oggi, nel mese di febbraio, a seguito dell'inadempienza del recepimento nei termini della legge comunitaria precedente, possano

da come si può vincere dagli emendamenti presentati e dalla discussione in Commissione finanze, nulla è stato concesso alle opposizioni per intervenire e modificare questo provvedimento, così urgente e così immutabile, pur con delle migliorie possibili e necessarie

L'Aula del Senato, a fronte di questa erronea - a mio avviso - urgenza, addirittura non è neanche in potestà di apportare le modifiche pur necessarie, anche se contenute, che in Commissione finanze avevamo proposto. proposto. Se tanta e tale deve essere la dirittura di considerazione delle norme che sono all'interno di questo decreto, ebbene, facciamo allora questa opera di grande correttezza, ma facciamola fino in fondo, non solamente nella parte che può interessare. Stiamo bene attenti la procedura del decreto per l'assorbimento nella normativa nazionale delle direttive delle Comunità;

- norme in recepimento che non hanno carattere di urgenza (come richiamato invece dalla legge n. 11 del 2005 e dalla Costituzione), creerebbe, anche con lo strumento della ricezione nella nostra normativa delle norme di diritto europeo, un ulteriore spazio di illegittimità, con l'inserimento di norme che invece dovrebbero dovrebbero essere valutate nella sede opportuna. Tale sede, per quanto riguarda le Camere, è la legge comunitaria. Ritengo, pertanto, signor Presidente,

stralciato, non potremmo che essere d'accordo sulla costituzionalità del provvedimento nel suo insieme. La questione rimane tuttavia fondata e, per questo motivo, auspico che l'Aula la approvi e che venga quindi rinviato in Commissione

Ne ha facoltà. VILLONE *(Ulivo)*. Signor Presidente, ho ascoltato con tutta l'attenzione possibile l'illustrazione della pregiudiziale, di cui, purtroppo, non ho avuto modo di leggere il testo. Mi pare di aver capito, però, che dal punto di vista strettamente costituzionalistico - che è quello che ci riguarda - il collega che ha svolto l'illustrazione ha richiamato la disciplina che viene posta sull'iniziativa di Governo quanto all'attuazione di norme comunitarie da parte della cosiddetta legge comunitaria, cioè da parte della legge che disciplina in via generale l'introduzione delle normative comunitarie nel nostro sistema. Indiscutibilmente questa normativa esiste, ma va letta, io credo, come dicono i tecnici, *secundum* *Constitutionem*, perché nella lettura che ne dà il collega che mi ha preceduto sicuramente ci sarebbero profili di incostituzionalità. Infatti, il collega sembra ritenere che quella disciplina possa precludere l'iniziativa governativa di attuare la disciplina comunitaria con l'utilizzazione di uno strumento di urgenza qual è il decreto-legge. A questo proposito mi permetto di dire che la legge ordinaria, che disciplina in termini generali l'introduzione nel nostro sistema della normativa comunitaria, non può ovviamente porre limiti insuperabili ad una facoltà che è sancita direttamente in Costituzione per il Governo. il potere di iniziativa legislativa, anche per quanto riguarda i decreti-legge, non perché glielo attribuisce la legge ordinaria, ma perché glielo affida direttamente la Costituzione.

la presentazione di un decreto-legge da parte del Governo, qualora questo ritenesse che ne esistono le condizioni, e cioè i presupposti costituzionali di necessità e di urgenza. Quella normativa, quindi, deve essere letta come una regola che in termini generali detta le modalità per la presentazione da parte del Governo di atti che introducono la normativa comunitaria nel nostro sistema, ma non ini termini che escludono l'esercizio di facoltà direttamente proprie del Governo quanto all'adozione di quegli atti. La domanda che dobbiamo porci quando ci troviamo di fronte all'adozione di un decreto‑legge,

E da questo punto di vista credo che la risposta l'abbiamo compiutamente avuta nella relazione del senatore D'Amico, il quale ha ampiamente illustrato le condizioni di necessità e di urgenza che sorreggono l'adozione del decreto, per quanto mi riguarda conclusivamente illustrato. In sostanza, il collega D'Amico in maniera molto ampia ed esauriente, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa alle banche e al sistema finanziario,

a prese di posizione della Comunità europea, ma proprio in condizioni di svantaggio competitivo, con danno per il nostro Paese. Questo ho colto come nocciolo più significativo, di sostanza, al di là delle

il riconoscimento della necessità ed urgenza. In secondo luogo, il relatore ha ampiamente richiamato le prese di posizione dell'Unione Europea, che su questo particolare profilo del sistema bancario e creditizio, e anche sugli altri toccati successivamente nei vari articoli di questo decreto, sono connesse a specifiche tematiche che l'Unione Europea in generale e persino la Corte di giustizia hanno assunto a base di proprie determinazioni. Quindi, anche da questo secondo punto di vista non pare discutibile che l'urgenza e la necessità vi sia, per la decorrenza del tempo che di per sé pone il nostro Paese in difficoltà di fronte all'Unione Europea, tra l'altro per taluni versi con procedure di infrazione già in atto. Abbiamo pertanto a disposizione un ampio insieme di considerazioni che ci fanno ritenere che, nella specie, questo decreto sia ampiamente supportato quanto all'esistenza dei presupposti di necessità ed urgenza nella situazione che il Governo ha preso in considerazione nella scelta di adottare questo particolare strumento normativo. Né, per le ragioni che dicevo prima, può essere assunta in modo ostativo e in termini conclusivi l'esistenza di norme di legge ordinaria che, se fossero lette nei termini di poter impedire insuperabilmente al Governo di adottare lo strumento normativo in questione e, in genere, di esercitare facoltà che allo stesso Governo sono assegnate dalla Costituzione, non potrebbero che essere di per sé incostituzionali. Quindi, tale lettura non è possibile: una lettura, come dicevo, *secundum Constitutionem* ci dice che in questo caso è ammessa l'utilizzazione dello strumento di urgenza, né potrebbe essere impedita da una legge ordinaria che volesse leggersi in senso contrario. Pertanto, a mio avviso, viene meno il fondamento determinante che veniva assunto dal collega che mi ha preceduto e dunque si rende manifesto che la questione pregiudiziale deve essere respinta.

quanto con molta dottrina detto dal collega Villone rappresenta una risposta sufficiente, ma la relazione del collega D'Amico motiva motiva ampiamente le ragioni di necessità e di urgenza, non solo per gli articoli 1 e 2, che peraltro vengono riconosciute dello stesso senatore Franco come meritevoli della valutazione di urgenza e indifferibilità per cui il decreto risulta ampiamente motivato. Il semplice fatto che vi sia peraltro una sorta di incidente, di incidente, nel senso che vi è un articolo 3 che è stato soppresso (lo ricordava il collega D'Amico) in sede di discussione alla Camera dei deputati perché è intervenuta nel frattempo una normativa che ha risolto il problema relativo all'organizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti; conferma, se ce ne fosse bisogno, che la scelta del Governo di intervenire con un decreto

rivolta a recepire la normativa comunitaria in base alla quale abrogare il provvedimento in materia di deroga alle

ai fini della efficacia dell'intervento del Governo sulla norma regionale, l'altra ai fini del recepimento utile e non differito dei finanziamenti dell'Unione Europea a favore dei giovani e dei programmi a sostegno delle attività giovanili nel nostro Paese, il ricorso al il ricorso al decreto. In sede di discussione, magari, ci soffermeremo ulteriormente sui singoli punti

come si fa a non riconoscere l'urgenza di misure che, recependo le norme di Basilea 2, intervengono a modificare, rafforzare e qualificare gli interventi di controllo sul sistema creditizio e finanziario del nostro Paese, in funzione di renderlo più trasparente, più efficiente e più efficace e quindi più funzionale a una politica di crescita e sviluppo? Bisognava aspettare la scadenza

va bene che è martedì grasso e forse siete eccitati per questo, ma i colleghi stanno intervenendo sulla questione pregiudiziale e quindi si prega di mantenere un minimo di rispetto. Prego, senatore Ripamonti. Presidente, ovviamente, interverrò solo sulla parte relativa alla sussistenza dei requisiti di costituzionalità,

per recepire alcune norme e direttive di carattere comunitario. In particolare ricordo, Presidente, che i primi due articoli intervengono sul Testo unico bancario e su quello di intermediazione finanziaria e recepiscono gli Accordi di Basilea. Ovviamente, nel merito vi sarebbe molto da dire riguardo a come ciò incida

il provvedimento interviene su questa materia sapendo che il termine di recepimento della direttiva scadeva il 31 dicembre e, di conseguenza, ritengo vi fosse la necessità di utilizzare

concernenti anche il sistema dell'informazione e della maggior trasparenza rispetto ai consumatori, che hanno subito in questi anni danni rilevanti nel loro rapporto con il sistema creditizio a seguito dei *crack* finanziari,

rilevanti, sulle quali a mio parere c'è necessità di intervenire in modo urgente. Mi riferisco all'articolo 4, in particolare laddove si provvede all'esecuzione di una ordinanza della Corte di giustizia europea del 2006, che chiede

specie cacciabili. È una questione rilevante sulla quale bisognava intervenire - ripeto - con estrema urgenza, anche perché, forse dal punto di vista

della legislazione comunitaria, queste sono norme di rilevanza decisiva, soprattutto quando si tratta di rispettare alcune regole. Infine, l'articolo 5 interviene sull'istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani e per l'assegnazione delle risorse finanziarie e per il suo funzionamento. Ritengo questa una materia importante, che necessita appunto di intervenire in modo urgente, per dare attuazione alla decisione

dell'attenzione da parte del nostro Governo di intervenire in modo celere su queste materie, dando risposta ai problemi che i settori giovanili hanno anche nel nostro Paese ed attuazione ad una direttiva comunitaria molto precisa al riguardo. Per questi motivi ritengo che

faccio mie le valutazioni del collega Franco Paolo, che ha esposto notevoli dubbi di presenza dei requisiti d'urgenza, quindi di compatibilità costituzionale di questa norma nel contesto della disciplina dei rapporti tra il nostro Paese e la Comunità Europea e la necessità di adeguare il nostro ordinamento alla normativa europea. Credo sia significativo che l'articolo 5 preveda una norma di tal genere, eccezionale nel panorama dell'adeguamento dell'ordinamento italiano all'ordinamento comunitario. Non so se vi sono precedenti di ricorso a decreti-legge per adeguare l'ordinamento a direttive comunitarie non scadute e in questo caso - possiamo dire - fresche di stampa,

e quando naturalmente vi erano tutti i tempi sufficienti per seguire le procedure previste dalla legge La Pergola aggiornata alla riforma del Titolo V della Costituzione. però, Presidente, è un'occasione per reintrodurre in Aula un tema che credo debba formare oggetto di riflessione da parte di tutti i soggetti che intervengono nel processo legislativo. Abbiamo una serie di norme non solo di rango costituzionale, ma di legge ordinaria, sia nei contenuti che nelle procedure, che vincolano il legislatore. ci dicono che in alcune materie occorre fare così; vi sono altre norme che dicono che in altre materie occorre procedere così.

introdurrà novità nel nostro ordinamento e sarà difficile far valere le leggi anteriori che vincolano il legislatore, salvo ricorso alla Corte costituzionale. Tuttavia, le norme che abbiamo introdotto in molte leggi che definirei di rango costituzionale, ad esempio la legge sulla contabilità,

Esse vincolano altresì il Governo nel momento in cui approva un decreto-legge; vincolano il Presidente della Repubblica nel momento in cui è chiamato a promulgare una legge e vincolano una Camera, sia il Senato che la Camera dei deputati, nel momento in cui porta avanti una determinata procedura. Se non entriamo in quest'ordine di idee, non potremo mai dare valore e vigore a norme sulle quali magari vi è

di rango istituzionale e di rango politico superiore, quasi paracostituzionale, affidando poi la violazione di quei precetti a leggi approvate che sono il frutto di un confronto politico basato su numeri di maggioranza e opposizione spesso dettate dalla contingenza e dal momento politico. Se non acquisiamo tale cultura e non cerchiamo di sforzarci di tradurre questi principi in regole per il nostro comportamento e per il comportamento degli altri soggetti coinvolti nel processo legislativo, possiamo ben parlare di valore istituzionale, di valore superiore, di valore che travalica le contrapposizioni politiche di un provvedimento rispetto a un altro, ma non avremo dato nessun contenuto vero ai nostri propositi. La legge comunitaria, che con tale articolo viene sostanzialmente derogata, ha valore costituzionale e quindi ritengo estremamente grave

Il provvedimento d'urgenza che oggi è al nostro esame contiene disposizioni certamente munite dei requisiti di legge e corrisponde quindi ai presupposti di necessità e urgenza prescritti dalla Costituzione. Tali requisiti si evincono chiaramente nella parte prevalente del testo normativo che dispone il recepimento di due direttive comunitarie (2006/48/CE e 2006/49/CE), comportando modifiche al Testo unico in materia bancaria e creditizia e al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria. Vi sono, inoltre, una misura conseguente a una pronuncia giurisdizionale comunitaria riferita a una legge regionale della Liguria e altre che, rispettivamente, istituiscono, ancora in attuazione di una

Urgenza e necessità, dunque, si evincono dal merito del testo sinteticamente appena esposto e altresì dalle ragioni di opportunità improcrastinabili nel recepimento di norme comunitarie che impongono il ricorso alla decretazione d'urgenza.

che rappresentano la parte caratterizzante del provvedimento in questione, è uno stimolo assai rilevante per la modernizzazione del nostro sistema bancario e del nostro sistema economico. In particolare, il decreto-legge apporta numerose modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, soprattutto con riferimento all'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle banche, sugli istituti di moneta elettronica e sui gruppi bancari, nonché sulle convergenze internazionali della misurazione del capitale e dei requisiti patrimoniali per la vigilanza bancaria. Gli interventi legislativi sono, tuttavia, contenuti nei limiti minimi necessari per l'estensione dei poteri regolamentari e di vigilanza, coerentemente con la logica del TUB, che rimette le prescrizioni di carattere tecnico ad atti regolamentari delle autorità creditizie. L'obiettivo che ci si propone è quello di assicurare, con una gestione trasparente del credito, una stabilità al sistema bancario, ma in funzione del rafforzamento e della competitività dell'intero sistema economico, che oggi ha continua necessità di capitali per investire in ricerca e sviluppo e aumentare la capacità di innovazione. Inoltre, punta a determinare un legame del tutto diverso tra banca e impresa, fondato su fiducia reciproca e supportato da informazioni reali e continuamente aggiornate, vincolate all'effettiva capacità di produrre reddito anche nella prospettiva di una crescita futura e non solo per obiettivi a breve termine. Credo si possa convenire sul fatto che proprio il sistema economico italiano, in particolare, ha bisogno di una maggiore intersezione tra banche, imprese e risparmiatori per dischiudere molte delle sue potenzialità. Il maggior valore di questa normativa è il realismo delle analisi nel rapporto rischio‑redditività e la necessità di aggiornarle di continuo seguendo dunque le aziende e il mercato molto più da vicino. Ciò consente di affrontare meglio e con maggiori strumenti anche l'esigenza di sostenere in investimenti, in innovazione e in ricerca, che sono i più rischiosi, ma possono generare maggior reddito nel futuro e maggior crescita economica. L'atteggiamento che le banche sono chiamate a sviluppare va dunque in direzione di una maggiore responsabilità, sia nei confronti delle aziende, sia nei confronti dei risparmiatori. Certo, per le banche si avrà una maggior discrezionalità nelle decisioni imprenditoriali di quelle imprese che chiedono un credito: in questo senso, la banca, attraverso l'uso di *rating* interni e di *rating* esterni, e dunque grazie a una maggiore flessibilità nella misurazione del rischio di credito rispetto ai criteri più meccanicistici in precedenza vigenti, diventa una sorta di consulente‑controllore di qualità dell'impresa. Ma se l'impresa è solida, i suoi progetti validi, e le prospettive di remunerazione dell'investimento affidabili, anche l'impresa ne trae vantaggio perché meno la banca rischia, meno ha necessità di accantonare denaro per tutelarsi, meno lo deve ricaricare sui clienti. Il recepimento del nuovo Accordo di Basilea, pur conseguendo l'obiettivo di armonizzare la normativa su scala globale, viene realizzato, con il provvedimento che discutiamo, in modo da creare una convergenza sostanziale sul piano prudenziale, ma senza appiattire su un modello unico le tecniche operative e contrattuali e, di conseguenza, senza creare situazioni di svantaggio competitivo per il nostro Paese. In particolare, va sottolineata per importanza la parte di modifiche per dotare le autorità di vigilanza (segnatamente la Banca d'Italia) dei necessari poteri, non solo relativamente al rischio del credito, ma anche del cambio e dell'interesse, nonché circa l'obbligo di informazione al mercato perché la clientela possa scegliere gli istituti più affidabili. Indubbiamente stiamo parlando di un processo che, per il suo pieno sviluppo, dovrà scontare una fase di messa a regime, e di crescita culturale e professionale, sia da parte dei diversi più affidabili. Indubbiamente stiamo parlando di un processo che, per il suo pieno sviluppo, dovrà scontare una fase di messa a regime, e di crescita culturale e professionale, sia da parte dei diversi istituti bancari sia da parte del mondo delle imprese. Le nuove regole non realizzano soltanto un significativo progresso nei livelli di sicurezza e stabilità dei sistemi bancari, ma ottengono anche il risultato di accrescere la libertà di scelta degli intermediari e i vantaggi economici ricavabili da miglioramenti dei sistemi di gestione dei rischi. In conclusione, ci si mette in una prospettiva che sollecita l'efficienza delle banche e l'efficienza del sistema creditizio del nostro Paese. Sono premiate con minori obblighi di capitale quelle banche, grandi e piccole, che utilizzano metodi di quantificazione più precisi e più efficaci nella gestione dei rischi di credito. In questo senso, il recepimento dell'accordo rappresenta anche un fattore di selezione perché accentuerà la concorrenza restituendo quote di mercato. Nell'ottica dell'attuazione di Basilea 2, da molte parti si sono avanzate preoccupazioni circa le ricadute sul sistema delle piccole e medie imprese italiane, perché le piccole e medie imprese possono avere minori possibilità di generare reddito o di generarne di ingente; inoltre, sono solitamente a conduzione familiare e quindi refrattarie all'ingresso di soci e capitali esterni e a volte anche non attrezzate nel settore analisi e gestione della finanza. La conseguenza è che le piccole e medie imprese in Italia risultano avere un livello di capitalizzazione basso rispetto, per esempio, alle consorelle francesi, britanniche o alle imprese tedesche. È proprio a partire da questa situazione di criticità che è importante mettere in evidenza anche tutta la potenzialità di un cambiamento così forte come quello che può essere innescato dal provvedimento che noi discutiamo. Perché tante piccole e medie imprese costituiscono in molti casi centri di eccellenza che operano su mercati a livello internazionale e hanno bisogno, confrontandosi con quei mercati, di essere sostenute da *partner* finanziari che si muovono in prospettive internazionali. In quest'ottica, il passaggio dalla figura della banca che presta denaro a quello della banca assistente, controllore e consulente, può certamente contribuire alla crescita delle piccole realtà in realtà più grandi e competitive. Non solo, ma anche con riferimento alla generalità della piccola impresa diffusa e alle sue esigenze di tutela, va evidenziata l'opera intelligente con cui nel provvedimento si è ricercato un adattamento alle specifiche esigenze

il riconoscimento della minore rischiosità dei prestiti assistiti da questa forma di garanzia, sia nelle opzioni regolamentari più semplici, che riguardano le banche minori, sia in quelle più complesse, utilizzate dalle grandi banche. La nuova disciplina, rispetto a Basilea 1, innova sensibilmente proprio e in particolare sulla capacità dei consorzi fidi di svolgere un ruolo di strumenti di mitigazione del rischio creditizio per le banche finanziatrici. Questa disposizione è destinata, anche per effetto della circolare di recente emanata in merito dalla Banca d'Italia, a produrre innovazioni significative. Penso, ad esempio, al processo di aggregazione delle tante cooperative artigiane di garanzia in consorzi di garanzia fidi di più grandi dimensioni. Un processo che risulta già avviato in Toscana, ad esempio, e ugualmente diffuso in Emilia, dove, anche sulla base di ricerche e valutazioni che sono attualmente in corso, si potrebbe pervenire a strutture su base regionale - questa è la tendenza a cui si lavorerà con ben altro profilo di solidità e incisività proprio a sostegno del sistema della piccola e media impresa: ed esperienze simili sono ormai in gestazione in tutto il Paese. Si tratta, attraverso lo strumento che veniamo ad approvare, di favorire un processo di enorme prospettiva, proprio nell'ottica del sostegno alle piccole e medie imprese, soprattutto quelle più giovani e più innovative. Signor Presidente, mi sono soffermato sugli aspetti di merito connessi al provvedimento, perché è su questo che mi auguro si concentri il dibattito, come è stato, almeno per una parte della discussione in Commissione (penso in particolare agli interventi dei colleghi Eufemi e Curto). Ovviamente non mi nascondo che abbiamo dovuto lavorare in tempi stretti e che proprio il presidente Benvenuto ha raccomandato al rappresentante del Governo che per i prossimi provvedimenti in materia, che sappiamo *in* *itinere*, si possa avere in Commissione maggior agio di discussione e più spazio per un nostro miglior concorso nella definizione degli stessi provvedimenti. Tuttavia, il tempo per un ampio dibattito - mi avvio a concludere è stato trovato, così come si è avuta una disamina di merito sugli emendamenti presentati: se c'è disappunto da parte dei colleghi dell'opposizione perché non sono stati accolti quegli emendamenti, non si può però accusare la maggioranza di comportamento arrogante e di indisponibilità al dialogo. Il filo di un dialogo che noi cerchiamo sempre, spesso trovandolo - voglio darne atto - nell'interlocuzione informale, ma che poi si spezza, quando si arriva al momento dell'espressione di voto. Non so se oggi cambieranno gli atteggiamenti dopo la discussione generale in Aula; penso che, se questo non avverrà, si sarà persa una buona occasione - e me ne rammarico - per condividere insieme, anche con le opposizioni, un atto importante

siamo chiamati ad adempiere ad obblighi comunitari ai quali non era possibile ottemperare con lo strumento della legge comunitaria annuale. Sottolineo, in modo particolare, l'articolo 5 del disegno di legge n. 1299, che istituisce l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede a Roma, trasferendo ad essa le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventù, già costituita presso il Ministero della solidarietà sociale, che viene conseguentemente soppressa. Per l'attuazione di tale nuova struttura viene autorizzata la spesa di 600.000 euro annui per il triennio 2007-2009. Anche questa, cari colleghi, è una ragione di urgenza, perché, altrimenti, anche queste risorse potrebbero essere perdute. Il rilievo di questo passaggio è del tutto evidente: noi apparteniamo all'Unione Europea nella misura in cui realizziamo con gli altri Paesi dell'Unione i medesimi obiettivi, le stesse linee di azione e anche i medesimi strumenti, come appunto l'Agenzia in questione. Già il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 1719 del 15 novembre 2006, che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013. L'Agenzia è uno strumento per realizzare l'obiettivo fondamentale dell'Unione: rendere i giovani protagonisti, in ciascun Paese e in tutta l'Unione. Si tratta di favorire la loro iniziativa e il loro pieno inserimento nel tessuto sociale, culturale, politico dell'Unione, ben sapendo che il trattato sull'Unione Europea è fondato sui princìpi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la parità tra donne e uomini, la non discriminazione. Solo la promozione della cittadinanza attiva dei giovani può contribuire allo sviluppo di questi valori: essi vivranno in futuro se saranno posseduti dalla coscienza delle nuove generazioni. Questo - parlo per i mesi attuali della vicenda del processo europeo - è un passaggio storico per l'Unione. L'euro e l'allargamento, che già hanno effetti strategici per il futuro delle nostre società, attendono il completamento del Trattato costituzionale. Qui i popoli dell'Europa possono riconoscere il proprio destino futuro e sentire una più forte appartenenza al grande sogno europeo. È chiaro che tutto ciò è consegnato innanzi tutto alle nuove generazioni. Il programma «Gioventù in azione», che è iniziato il 1° gennaio 2007 e si concluderà il 31 dicembre 2013, abbraccia l'arco temporale di questa fase decisiva per l'Unione. Il programma è assai ricco e l'Agenzia nazionale non potrà che esserne un utile strumento per promuovere la cittadinanza dei giovani (e qui si intendono coloro che vanno dai 15 ai 28 anni); per sviluppare solidarietà e comprensione reciproca tra i giovani dei diversi Paesi; per accrescere lo sviluppo delle attività dei giovani nelle organizzazioni della società civile; per favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù; per sviluppare la partecipazione giovanile alla vita democratica dell'Unione; per incoraggiarne lo spirito di iniziativa; per favorire i giovani con minori opportunità o con disabilità; per incoraggiare la mobilità, lo scambio di buone pratiche; e per sostenere la cooperazione con i giovani del mondo, con i Paesi del vicinato dell'Unione Europea, come i Balcani. Solo tenendo fermo il quadro di riferimento posto dall'Unione si può comprendere il senso dell'Agenzia nazionale per i giovani. Signor Presidente, vorrei che fosse raccolta una raccomandazione: l'Agenzia è «per» i giovani, ma deve essere soprattutto «dei» giovani. È stato approvato alla Camera un emendamento aggiuntivo al comma 2 dell'articolo 5 assai utile; «le risorse dell'Agenzia» sono «prevalentemente utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali alla stessa attribuite» (è chiaro che l'esperienza ci mette in guardia dal rischio che poi le risorse servano per autoconservare lo strumento, anziché per promuovere il protagonismo dei soggetti a cui è rivolto). Quindi, non si sovraccarichi di burocrazia ciò che dev'essere invece tutto volto al protagonismo dei giovani. Le funzioni di indirizzo e di vigilanza, esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche giovanili e dal Ministro della solidarietà sociale sono un impegno forte in questa direzione. Anzi, è quanto mai opportuno che le stesse politiche giovanili in Italia assumano quanto più è possibile un profilo europeo e internazionale, perché è proprio questo il mondo in cui la gioventù oggi vive: il mondo dell'incontro, del dialogo, del confronto;

*(Ulivo)*. Signor Presidente, mi permetta di far osservare che la conversione in legge del decreto-legge n. 297 del 2006, i cui contenuti sono stati pregevolmente e compiutamente illustrati dal relatore, giunge all'attenzione dell'Aula dopo un approfondito esame svoltosi in Commissione, anche in relazione alle modificazioni apportate al testo originario dalla Camera dei deputati. Un esame - dicevo - approfondito, esteso e partecipato, sui vari aspetti del provvedimento, pur nei tempi ristretti concessi dall' agenda dei lavori. Ritengo, quindi, abbastanza immotivata, sia sul piano politico che sul piano tecnico, la posizione assunta dalle forze di opposizione all'atto del voto finale con la scelta di abbandonare i lavori della Commissione competente. Credo ed auspico che la discussione in Aula potrà offrire l'occasione per ripianare i contrasti registratisi in quel frangente, anche tenendo conto della volontà mostrata dalle forze di maggioranza nell'aver raccolto, sotto forma di ordini del giorno, alcuni precisi contenuti di merito emersi nel corso del confronto in Commissione e proposti proprio dalle forze di opposizione. D'altra parte, come ribadito già dal relatore e da altri colleghi che mi hanno preceduto, il provvedimento alla nostra attenzione si caratterizza per un contenuto prevalentemente tecnico. Si tratta, infatti, di disposizioni per le quali, appunto, sussistono effettivamente le ragioni di necessità e urgenza ai fini di una tempestiva introduzione nell'ordinamento giuridico italiano di significative norme e decisioni comunitarie. Anch' io voglio ricordare che con il testo all'attenzione dell'Aula si attua, in via prioritaria, il recepimento dei contenuti dell'Accordo del Comitato di Basilea sull'adeguatezza patrimoniale delle banche; ma si provvede, altresì a dare esecuzione, nell'articolo 4, all'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla sospensione dell'applicazione della legge della Regione Liguria n. 36 del 2006; e ancora, nell'articolo 5, si provvede a costituire l'Agenzia nazionale per i giovani, in attuazione della decisione n. 1719 del 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Si tratta a ben vedere di disposizioni, anche in questi casi, particolarmente urgenti e significative, che non possono essere ulteriormente dilazionate. Si è detto del particolare significato delle disposizioni alla nostra attenzione soprattutto per quanto riguarda i contenuti degli articoli 1 e 2 del decreto. Qui, del resto ricordava il relatore), si colloca il «nocciolo duro» del provvedimento ed è su questa parte in particolare che si è svolta l'ampia discussione in Commissione, Con gli articoli 1 e 2 si provvede, infatti, al recepimento degli Accordi cosiddetti di Basilea 2. Si tratta di una normativa che parla direttamente al nostro intero sistema economico e produttivo, chiamando la struttura bancaria del Paese ad assumere più precise responsabilità. Obiettivo prioritario di Basilea 2 è, infatti, quello di determinare un legame più stretto tra la solidità patrimoniale delle banche e la richiesta dei finanziamenti, attraverso l'utilizzo di *rating* interni ed esterni. Sono tre i punti fondamentali che distinguono l'Accordo di Basilea 2 e che ritengo opportuno qui richiamare: le regole sui requisiti minimi di capitale per le imprese bancarie, la disciplina della vigilanza, l'utilizzo - appunto - dei *rating* interni ed esterni per la valutazione del rischio di credito. Tali criteri offrono la possibilità di superare le difficoltà emerse rispetto a quelli dettati nel precedente Accordo di Basilea, proprio in ragione del loro carattere di maggiore flessibilità. In particolare, quindi, ritengo opportuno far osservare che, per quanto riguarda i requisiti minimi di capitale, viene certamente adottato un parametro analogo a quello previgente, ma che in ogni caso consente una maggiore elasticità nella misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali. E, ancora, degna di nota risulta essere la scelta di attribuire alle banche centrali, ovvero alla Banca d'Italia, nel nostro caso, poteri regolatori in merito alla valutazione del rischio di credito e di adeguatezza patrimoniale. Altrettanto meritevole d'attenzione è la messa in atto di giudizi di *rating* da parte di banche e agenzie ufficiali che può aiutare la crescita del mercato, così come l'attuazione di strumenti e misure volte alla trasparenza delle informazioni al pubblico.

senza dubbio il sistema bancario del Paese e lo stesso sistema produttivo è chiamato a confrontarsi con criteri di omogeneizzazione già, peraltro, in vigore in altri Paesi, spesso con noi anche in dura competizione. È vero in ogni caso - tendo a ribadirlo che le disposizioni in esame volgono sicuramente lo sguardo verso un ulteriore passo per la modernizzazione del nostro sistema economico, e di quello bancario in particolare. D'altra parte, va segnalato lo sforzo che le norme in esame attuano nella realizzazione di una integrazione della normativa generale con le peculiarità del nostro sistema economico e produttivo. A tal proposito, anch'io voglio segnalare all'attenzione del nostro confronto il fatto che si è teso a rendere possibile il riconoscimento della minore pericolosità dei prestiti assistiti dalle forme di garanzia offerte dai consorzi fidi. Rispetto all'Accordo di Basilea 1, dunque, si provvede ad una innovazione di sostanza, riconoscendo ai consorzi fidi la capacità di fungere da strumenti di integrazione del rischio creditizio per le banche finanziatrici. Queste sono alcune delle motivazioni e degli argomenti che portano a considerare la conversione in legge del decreto in esame come un adempimento opportuno e necessario, al fine - io credo - di rendere sempre più competitive le imprese bancarie nei mercati internazionali. L'ottimale utilizzo e allocazione dei capitali finanziari potrà rendere inoltre, a mio avviso, più solido il nostro sistema economico in tutte le sue particolarità e le sue articolazioni.

il Presidente del Senato, senatore Marini, ha consentito l'opportunità di chiarire uno sgradito episodio accaduto in Commissione finanze e tesoro, nella seduta notturna di mercoledì scorso, con all'ordine del giorno proprio il decreto-legge al nostro esame. Chiarimento che mi auguro abbia ricondotto nel reciproco rispetto i rapporti fra maggioranza e opposizione. Circa il provvedimento al nostro esame, ravvisiamo una costante nelle modalità e tempismo dei Governi in carica circa le direttive comunitarie che vengono proposte al Parlamento nella cosiddetta legge comunitaria, legge che spesso si trascina durante l'arco di un anno da una Camera all'altra e diventa il tramite legislativo sul quale introdurre nuove tematiche, così come stava per accadere in prima lettura alla Camera dei deputati sul provvedimento al nostro esame. Infatti, dal testo del decreto-legge concernente il recepimento di due direttive comunitarie, in quell'Assemblea è stato espunto l'articolo 3 in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti ed è stato dichiarato inammissibile un emendamento del Governo che andava a modificare la legge sugli immigrati, la cosiddetta Bossi-Fini.

I correttivi apportati al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle banche, sugli istituti di moneta elettronica e sui gruppi bancari, oltre che sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei requisiti patrimoniali per la vigilanza bancaria, derivano dall'Accordo del Comitato di Basilea del 25 giugno 2004 che è la fonte della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, in data 14 giugno 2006, concernente l'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio. gli articoli 1 e 2 caratterizzano il provvedimento, che è complesso e di notevole tecnicalità: basta far riferimento alla disciplina sulla prassi di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito fondato sui *rating* interni, sul trattamento prudenziale delle tecniche per la riduzione del rischio di credito e delle cartolarizzazioni e sul calcolo dei requisiti patrimoniali minimi del rischio operativo. evidente che le vicende bancarie di questo ultimo decennio hanno prodotto crisi non indifferenti circa l'adeguatezza patrimoniale e la trasparenza del rapporto fra banche e impresa, e hanno indotto il legislatore comunitario ad emanare nuove norme che regolano i requisiti minimi di capitale, il controllo prudenziale ed uno stringato coordinamento riguardo all'informazione al pubblico da richiedere alle banche. È quindi condivisibile la modifica del comma 10 dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che disciplina lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e tutte le autorità e soggetti esteri indicati nelle direttive comunitarie non più come facoltà, ma come prescrizione legislativa. Così pure le altre modifiche che disciplinano i poteri di vigilanza regolamentare della Banca d'Italia sulla adeguatezza patrimoniale con riferimento alla valutazione dei rischi utilizzando informative di società o enti esterni, sempre su disciplinari elaborati ed autorizzati dalla stessa Banca d'Italia. Non si comprende, invece, perché la facoltà di cui al citato comma 10 dell'articolo 7, tramutata in prescrizione, non sia stata estesa anche al rapporto con le banche nazionali, considerato che gli accadimenti in casa nostra inerenti ai *bond* argentini e ai *crack* della Parmalat e della Cirio sono esempi che alla stragrande maggioranza dei cittadini appaiono caduti nella banalizzazione di una ricerca di responsabilità rimpallata, laddove la palla è stranamente scomparsa. Di contro, non è accettabile che nel provvedimento sia stata inserita la norma che pone a carico del richiedente la valutazione del rischio d'impresa, invece di addebitarlo alle stesse banche. Vero è che il sistema bancario è impegnato da tempo nell'attuazione delle modifiche introdotte con la legge finanziaria 2005 del Governo Berlusconi, con un notevole sforzo (gliene diamo atto), che ha reso necessaria anche un'attenta opera di formazione del personale di sportello, impegnato nel delicato compito di acquisizione di dati sensibili da parte della clientela. Così come è noto che il decreto Bersani ha instaurato un rapporto tra banche e fisco con funzioni di per sé tipiche delle amministrazioni statali, in una dimensione pressoché sconosciuta negli altri Paesi dell'Unione. Comunque, signor Presidente, considerando la normativa in essere contenuta nel Testo unico delle leggi bancarie e il lavoro svolto dal Comitato di Basilea 2, siamo forzatamente d'accordo sulle due direttive, se non altro perché si fa riferimento alle competenze del Comitato, che è formato dai rappresentanti delle Banche centrali e delle autorità di vigilanza bancaria di numerosi Paesi, tra cui il nostro, ed anche perché esse sono imposte dall'appartenenza all'Unione Europea, così come accade, a maggior ragione, quando i provvedimenti dell'Unione Europea sono imposti da sentenza. Riteniamo, tuttavia, che nel compilare il presente provvedimento non si sia tenuto conto di alcune considerazioni di «sistema Paese» che riguardano l'Italia e che andavano fatte anche sulla base della formulazione delle stesse direttive, che consentono di far salvi i rispettivi ordinamenti nazionali, pur attraverso l'utilizzazione di princìpi comuni. Infatti, non possiamo ignorare che il nostro sistema bancario è antiquato proprio rispetto al rapporto creditizio, e non con la grande impresa, che ha risorse proprie, capitale tecnologico e manageriale all'avanguardia, facilità di accedere al mercato finanziario, attraverso l'emissione di titoli e obbligazioni, e al mercato del credito; ma nei confronti di quel mondo della piccola e media impresa che, se negli anni Settanta è stata la promotrice dei distretti industriali e del *Made* *in* *Italy*, salvando il nostro paese da una profonda crisi, oggi è asfittica sia nel capitale che, purtroppo, nella managerialità, spesso confusa da uomini carichi di esperienza e pragmaticità ai limiti del lecito, ma privi della conoscenza del sistema economico-finanziario che regola i rapporti che si instaurano con l'internazionalizzazione e la globalizzazione. Il ministro Bonino, che ha firmato il presente decreto, dovrebbe sapere che gli strumenti istituzionali (ICE, SACE, SIMEST), oltre che il sistema bancario, messi a disposizione della produzione nazionale, sono da tempo cristallizzati da un loro ordinamento travisato, che guarda che guarda all'interno della propria struttura più che dare un servizio all'utenza. E, sebbene in questi ultimi anni sia mutato lo scenario politico nazionale e si sia cercato di riguadagnare il tempo perduto, tuttavia ci troviamo nel mezzo di un processo evolutivo che ci costringe a dover rincorrere gli altri, emanando provvedimenti legislativi che risultano obsoleti il giorno dopo la loro entrata in vigore. Per dirla in breve, l'arte della furbizia e dell'arrangiarsi mal si adatta al mercato internazionale, che prevede una conoscenza del sistema Paese dove le banche debbono essere il sostrato su cui poggiare il proprio rischio di impresa. Questa era l'occasione, signori del Governo, ed ancora una volta ci siamo fermati a recepire quello che gli altri hanno deciso fuori dall'Italia; ci siamo accodati per l'ennesima volta ad una normativa condivisibile, ma fatta in casa d'altri per la casa d'altri. E, infine, prendiamo atto che nel presente decreto ci occupiamo di storni, uccelli dalle bellissime evoluzioni nei nostri cieli, con scarichi biologici non sempre accettabili sulle strade delle nostre città, e con qualche dubbio rileviamo che si sostituisce l'Agenzia nazionale gioventù con l'Agenzia nazionale per i giovani, corredandola di facoltà per le assunzioni di personale, con una quota di finanziamenti pari al doppio di quanto previsto nell'Unione e addirittura con un consiglio di amministrazione composto di otto membri, laddove tutto il personale dell'Agenzia annovera appena sedici dipendenti. C'è solo da augurarsi che questo organismo, che l'Unione impone come indipendente, rimanga tale e non diventi uno strumento politico per fini partitici. È davvero poco e, poiché il testo è palesemente blindato, voteremo contro questo provvedimento per insufficienza propositiva di questo Governo. *(Applausi

recependo alcune direttive dell'Unione Europea, ma Basilea 2 ha un significato internazionale di controllo del credito molto più ampio rispetto ai confini, pur estesi, dell'Unione Europea),

modificato, rivisto e aggiornato, soprattutto nel nostro Paese, che presenta una struttura della piccola e media impresa particolarmente diversa, rispetto agli altri Paesi interessati dalle norme di Basilea 2, e cioè dalle norme che danno attuazione alle direttive

indubbiamente con grande attenzione e capacità da parte delle attività imprenditoriali e delle attività finanziarie.

enti creditizi, elimina le differenze più rilevanti nella legislazione degli Stati membri, mira a salvaguardare il risparmio, crea condizioni di uguaglianza nella concorrenza tra le banche, rafforza il sistema bancario, fissa requisiti patrimoniali ben determinati. determinati. Questi aspetti sono stati correttamente illustrati dal relatore D'Amico e anche discussi in Commissione. La seconda direttiva, dovuta proprio al fatto che le imprese di investimento in queste condizioni corrono, per quanto riguarda il portafoglio di negoziazione, gli stessi rischi degli enti creditizi, fissa requisiti di adeguatezza patrimoniale che si applicano alle imprese di investimento e agli stessi enti creditizi. Da questo brevissimo sunto vediamo ovviamente che le norme non possono che essere ritenute assolutamente importanti e necessarie per il nostro Paese, nonché

devono corrispondere norme che permettano di avere criteri comuni, onde evitare che vi siano sistemi con livelli concorrenziali, chiamiamoli così, diversi.

dimostra che l'attenzione a questi temi anche da parte di chi oggi è all'opposizione c'è sempre stata ed è stata un'attenzione molto forte e determinata. Oggi ci troviamo comunque a recepire norme di direttive dell'Unione Europea che condividiamo,

a Basilea 2 un'interpretazione legata in maniera più stretta alle esigenze particolari della finanza, dell'industria, del sistema bancario del nostro Paese. Tutto ciò, però, non ci è stato concesso.

anch'essi vanno, pur trattando un argomento totalmente diverso, nella direzione di dare un contributo al provvedimento. Anche in questo caso, però, per le motivazioni più diverse, gli emendamenti dell'opposizione e della maggioranza sono stati rigettati.

ed incisive modificazioni al Testo unico delle leggi in materia creditizia e bancaria: maggiore sicurezza e stabilità dei sistemi bancari; nuove metodologie nei sistemi di valutazione e gestione dei rischi; più approfonditi controlli delle banche centrali, anche in ordine alla valutazione circa l'adeguata massa patrimoniale necessaria per l'esercizio dell'attività bancaria; maggiore disciplina del mercato e trasparenza (vengono introdotte nuove e più incisive regole di trasparenza per l'informazione al pubblico in ordine ai livelli patrimoniali, ai rischi e alla gestione dei rischi). Con l'articolo 1, lettera *a*), con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle banche, sugli istituti di moneta elettronica e sui gruppi bancari, nonché all'attuazione delle misure derivanti dall'Accordo di Basilea sulle nuove modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, basate anche sul metodo dei *rating* interni, viene prescritto che la Banca d'Italia scambi informazioni con tutte le le altre autorità e soggetti esteri indicati nelle direttive comunitarie, anche se diversi dalle autorità competenti degli Stati comunitari e degli altri Stati. In tal modo, viene ampliato il raggio dello scambio favorendo un maggiore flusso ed una maggiore trasparenza di informazioni. Ma, più di tutto, dall'applicazione di questa disciplina deriva l'obbligato presupposto di un elevato grado di convergenza dei criteri operativi e di cooperazione tra le autorità preposte, posto che le regole sui requisiti minimi di capitale e sul processo di controllo prudenziale dovranno essere applicate sia su base consolidata, sia alle filiazioni presenti in ciascun Paese. la lettera *b)* dell'articolo 1, all'Autorità di vigilanza è conferito il potere di disciplinare l'informativa che le banche debbono rendere al pubblico sull'adeguatezza patrimoniale, sul contenimento del rischio, sull'organizzazione amministrativa e contabile. Nel nuovo comma 2-*bis* viene statuito che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia debbano prevedere che ai fini della valutazione dei rischi le banche possano utilizzare sia le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, sia i sistemi interni di misurazione dei rischi. le misure che la Banca d'Italia può adottare nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti adottabili nei confronti di singole banche. Tali misure possono riguardare la restrizione delle attività o della struttura territoriale, come misura di vigilanza; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria; il divieto di distribuire utili o altri elementi del patrimonio. Con le modifiche introdotte alla lettera *c)*, viene infine ampliato il perimetro di esercizio della vigilanza su base consolidata. Al numero 1), modificando la definizione delle «società finanziarie», estendendo quindi la nozione fino a comprendervi le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, il servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento, nonché l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, ovvero la gestione del patrimonio di organismi d'investimento collettivo del risparmio di propria o altrui istituzione, mediante investimento in strumenti finanziari, creditizi o attraverso altri beni mobili o immobili. La nuova definizione di «società strumentali», contenuta nella lettera *c)* muta la precedente fattispecie di società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici. Con tale modifica viene precisato che la gestione di immobili può riferirsi all'esercizio della proprietà e dell'amministrazione degli stessi. Vengono modificate le definizioni rilevanti per la disciplina di vigilanza su base consolidata. Oggi, nella definizione di «società finanziarie» vengono incluse anche le società di gestione del risparmio. La nozione infatti viene estesa fino a comprendervi anche società che esercitano il servizio di gestione collettiva del risparmio, attraverso la formazione e l'organizzazione di fondi comuni di investimento, ovvero la gestione del patrimonio di organismi d'investimento collettivi del risparmio stesso. Con la lettera *d)* viene modificata la definizione «gruppo bancario». Infatti ora, con riferimento ai gruppi aventi come capogruppo una società finanziaria, ai fini dell'efficacia dei poteri di vigilanza da parte dell'Autorità nazionale, rileva il gruppo bancario composto dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali, che questa controlla. Con la lettera *f)* viene invece modificata la disposizione che determina quali siano i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata, escludendo le società finanziarie che hanno sede legale in un altro Stato comunitario e le altre società finanziarie diverse dalla capogruppo che controllano almeno una banca; di conseguenza, saranno soggette a vigilanza consolidata tutte le società che controllano almeno una banca. Con la lettera *g)* vengono modificati i poteri di vigilanza informativa della Banca d'Italia sui soggetti che fanno parte dei gruppi bancari. La nuova formulazione consentirà alla Banca d'Italia di applicare a determinati soggetti le norme sulla revisione contabile oggi previste per le società con azioni quotate; in tal modo, a tali soggetti, ancorché non quotati, potrà essere prescritta la revisione contabile da parte di una società di revisione. Verrà poi introdotto, attraverso questa normativa, l'obbligo per le società partecipate di fornire alla capogruppo le informazioni necessarie per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata. Con la lettera *h)* vengono modificati i poteri di vigilanza regolamentare della Banca d'Italia relativamente ai gruppi bancari mediante l'introduzione dell'obbligo d'informativa nei riguardi del pubblico e la possibilità di utilizzare valutazioni di rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, ovvero da sistemi interni di misurazione dei rischi. Con la lettera si permette alla Banca d'Italia di esercitare il potere di vigilanza ispettiva nei riguardi dei gruppi bancari. Essa potrà effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione di documenti e atti; potrà richiedere alle Autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i medesimi soggetti e potrà, inoltre, consentire che Autorità competenti di altri Stati comunitari partecipino alle ispezioni presso le capogruppo nel caso in cui queste abbiano società controllate sottoposte alla vigilanza delle medesime autorità. Con la lettera *l)* si innova in materia di collaborazione della Banca d'Italia con le Autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari agli effetti della vigilanza consolidata sui gruppi transnazionali. La nuova formulazione consentirà alla Banca d'Italia di concordare con le Autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione e ripartizione dei propri compiti ed esercitare la vigilanza consolidata. Il nuovo comma 1-*ter* stabilisce che, qualora la Banca d'Italia, nell'esercizio della vigilanza consolidata, verifichi l'esistenza di una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, sia tenuta ad informarne tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché - in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari - le competenti Autorità monetarie. Il presupposto per l'applicazione della norma è individuato in una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario. Con la lettera *m)* si interviene sugli intermediari finanziari, iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, introducendo gli obblighi di informativa in favore del pubblico. Alla lettera *n)* viene invece introdotto un nuovo articolo 116-*bis,* che disciplina la facoltà di disporre, sempre da parte della Banca d'Italia, che le banche e gli intermediari finanziari, autorizzati ad utilizzare sistemi interni di misurazione di rischi per la determinazione dei debiti patrimoniali, diano illustrazione dei fattori consolidati per la valutazione del merito di credito alle imprese che richiedono finanziamenti. Ecco, Presidente. Credo che l'illustrazione, seppure estremamente veloce, di una normativa che innova completamente, ancorché in attuazione, il nostro ordinamento in materia di controllo e di vigilanza della Banca d'Italia e di operatività delle società finanziarie che esercitano lo strumento creditizio sia per il nostro Paese, dopo tanti dibattiti politici, arrivato al traguardo finale con una norma eccellente che, per i motivi che ho appena sinteticamente accennato, ritengo di dover difendere e di cui chiedo l'approvazione in quest'Aula. PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà.

un coacervo di norme rappresentate unicamente dalla finalità e necessità di adempiere ad alcuni obblighi comunitari in scadenza o già scaduti. Si registra una sovrapposizione normativa con altre norme previste nella legge comunitaria, con duplicazioni in un caso e attribuzione di una delega contestualmente definita in altro decreto-legge. Cosicché si passa dal settore bancario e finanziario, come Basilea 2, alla assistenza a terra negli aeroporti, che rimane solo nel titolo, alla Agenzia nazionale dei giovani ed al prelievo venatorio. Abbiamo già rappresentato in Commissione finanze e poi in Aula la settimana scorsa il disagio delle opposizioni per un modo di procedere che riteniamo dannoso, così come il travolgimento degli strumenti di procedura offerti dalla legge n. 11 del 2005, la cosiddetta legge Buttiglione, implementanti dalla stessa. Come non si possono considerare prioritari i provvedimenti che riguardano Basilea 2, direttiva OPA, direttiva MiFID? Lo dico alla gentile senatrice Soliani, estensore del parere per la Commissione politiche dell'Unione. Tutto ciò dopo le vicende della scorsa settimana con il decreto di proroga termini, con modifiche operate attraverso emendamenti sul Patto di stabilità interno e sui *ticket* sanitari: quasi una minifinanziaria, attraverso, appunto, emendamenti, senza adeguata valutazione degli effetti finanziari. Non abbiamo sentito voci di indignazione rispetto alle coperture finanziarie, soprattutto nel disallineamento temporale, nella efficacia delle disposizioni. Tutto ciò mentre il Ministro dell'economia, nel suo candore, sollecita una riforma delle regole di bilancio, senza neppure tentare comportamenti nuovi ed adeguati, ma solo mosso dalla necessità di avere meno resistenze dalla sua contraddittoria maggioranza. Questo decreto è anche l'occasione per dimostrare la confusione legislativa che regna nella programmazione legislativa. Siamo stati costretti ad una corsa contro il tempo, con sedute anche notturne, per poi vedere spostato alla settimana successiva questo decreto. Identica cosa era avvenuta con la direttiva MiFID. In quel caso addirittura è stata pubblicata con grande ritardo sulla *Gazzetta Ufficiale*, non evitando il termine per l'esercizio della delega. E come non ricordare che in questo stesso provvedimento si fa riferimento pleonasticamante a quel CICR che si vuole abolire con la riforma delle Autorità di vigilanza, quelle stesse autorità che solo di recente, sul finire del 2006, venivano riprecisate nella loro articolazione specialistica dal Governo dopo il parere espresso dalle Commissioni parlamentari? Sappiamo bene come sono andate le cose. C'è stata Caserta. Quindi, da Prodi o da Bersani è venuto il «contrordine, compagni!», sconfessando platealmente il suo vice ministro Pinza. Per intanto si procede con super-Consob, soppressione di COVIP e ISVAP, cui avevate affidato il controllo sui prodotti previdenziali. Così come avete, con un atto di prevaricazione istituzionale, modificato, con un parere parlamentare, una norma sostanziale come il limite del 30 per cento nel possesso delle quote delle Fondazioni, ora vorreste addirittura utilizzare le norme di coordinamento finali o un ordine del giorno per modificare il titolo del presente disegno di legge di conversione del decreto-legge n. Dopo il brutto pasticcio della costituzione del fondo F21 e la relativa grancassa milanese, di cui si è naturalmente meravigliato il ministro Padoa-Schioppa (ma è stato lui ad andare a Milano con la sua batteria di Vice ministri, Sottosegretari e quant'altro), si comprendono bene le ragioni di questa scelta. Sarebbe una gravissima lesione al Senato se intervenisse un coordinamento finale su un testo nella sede sbagliata, perché in Senato, secondo la vostra posizione, non dovranno intervenire modifiche. Se vi erano correzioni da fare, occorreva farlo nella sede giusta e dunque alla Camera. Il decreto arriva in Aula con il parere obbligatorio della Commissione politiche dell'Unione, e dobbiamo dare atto al presidente Marini di essere intervenuto in questo senso, perché si disciplinano procedure di adeguamento normativo alla normativa comunitaria. Il Gruppo UDC si è mosso con spirito costruttivo soprattutto sulla direttiva concernente Basilea 2, che viene dopo un lungo percorso elaborativo che ha visto il coinvolgimento di soggetti diversi, stanti le ricadute sia sul versante delle imprese che delle banche. Abbiamo posto alcune questioni formali e sostanziali; abbiamo tentato di correggere macroscopici errori giuridico-formali; abbiamo registrato un atteggiamento di totale chiusura. Riteniamo che il Senato non possa essere solo il luogo della ratifica di decisioni prese in altre sedi, come ha riconosciuto (dobbiamo dire con sufficiente dovizia di particolari) il senatore Bonadonna. La stessa Conferenza delle Regioni ha evidenziato sull'articolo 4 di non condividere la fonte normativa dell'intervento urgente (articolo 120 della Costituzione) che prevede interventi sostitutivi da parte dello Stato nei confronti delle Regioni raccomandando che il caso non costituisca precedente e raccomandando un percorso istituzionale concordato. Si evince che volete evitare un confronto perfino con la Conferenza in cui avete una stragrande maggioranza. è poi il capolavoro dell'articolo 5, che vogliamo modificare perché rappresenta un gentile *cadeau* al ministro Ferrero. Queste funzioni di indirizzo delle politiche giovanili, prima esercitate dal Ministero del lavoro, non avvengono a costo zero. Infatti, non è chiaro quanta stima della spesa è già scontata e quanta sia pienamente riconducibile alle esigenze conseguenti alla creazione della nuova struttura. Troppo generico è il vincolo all'utilizzo delle risorse conseguenti ai nuovi oneri per il personale. A tal riguardo, il nostro Servizio studi ha fatto un lavoro egregio.

perché siamo preoccupati della presenza in ruoli istituzionali di ex partecipanti alla stagione degli anni di piombo. Era un modo per fare una cesura. E veniamo a Basilea 2. La direttiva guarda alla stabilità del settore bancario generando un legame nuovo tra banche e imprese. Essa si basa su tre pilastri: nuove modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza, controllo potenziale e disciplina del mercato. Cambiano i ruoli delle banche fra grandi e medio-piccole, perché focalizzate alla concessione di crediti alle piccole e medie industrie, valorizzando il localismo, dando attuazione ai princìpi di proporzionalità in relazione alle dimensioni, alle caratteristiche e alla rilevanza dei rischi e a un sistema di regole modulari nella misurazione e gestione dei rischi. Queste erano le nostre preoccupazioni. Si evita eccessiva prescrittività fornendo linee guida, presentando i vantaggi della regolamentazione, l'adattabilità alle innovazioni finanziarie e, soprattutto, libertà nella introduzione di tecniche di gestione. Le più forti preoccupazioni venivano proprio per il sistema delle piccole e medie italiane e tedesche che hanno le caratteristiche (soprattutto le imprese italiane) dell'impresa familiare, della bassa capitalizzazione e dei pluriaffidamenti bancari a breve. Sarà allora necessaria una ripartizione della funzione finanza all'interno delle imprese; la qualità del rapporto banca-impresa assumerà maggiore rilevanza. Si pone quindi il problema - come ho già sottolineato in Commissione - della definizione del livello della tassazione per le obbligazioni delle società, che va fissato al 12,50 Il Ministro dell'economia nei giorni scorsi ha dichiarato la guerra alle rendite. Ebbene, lo dimostri; non abbia eccessiva preoccupazione per le fondazioni bancarie ormai orientate verso il *profit;* guardi all'abbassamento del livello della tassazione delle obbligazioni delle piccole e medie imprese; ne sostenga la crescita, soprattutto nel quadro dei distretti e delle reti proiettate nella internazionalizzazione. Effetti per le imprese, dunque, che saranno interessate dalle nuove metodologie di determinazione del rischio che verrà valutato sulla base del rischio di credito e per le banche per il fabbisogno patrimoniale, che sarà minore quanto più le metodologie di valutazione del rischio saranno avanzate. Tutto ciò presuppone maggiore informazione, trasparenza e integrità. È positivo che il recepimento avviene senza appiattimento sul modello unico delle tecniche operative e contrattuali evitando situazioni di svantaggio competitivo. Basilea 2 sollecita l'efficienza delle banche, premiando quelle più efficaci nella gestione dei rischi. La Banca d'Italia sarà chiamata al compito delicato di convalidare i modelli di rischio utilizzati dalle banche ai fini di Basilea 2. Bene ha fatto l'Autorità di vigilanza ad emanare prontamente le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, in adesione ai princìpi della *better regulation*, di quelle tecniche e princìpi divenute obblighi normativi per la stessa autorità. La libertà di scelta impone agli organi aziendali la piena consapevolezza del sistema di gestione e del controllo dei rischi di cui si avvale. Richiede distinzioni di ruoli e di responsabilità. La scelta di un sistema di governo aziendale efficace assume valore di fattore competitivo determinante. Basilea 2 va vista dunque nel maggiore grado di libertà degli intermediari e nei vantaggi economici ottenibili dal miglioramento e nell'efficienza dei sistemi di gestione dei rischi. Tutto ciò implica decisioni complesse che si intrecciano con aspetti tecnici e di strategia. La questione Basilea 2 assume una rilevanza che non può essere però disgiunta dall'intero provvedimento, su cui esprimiamo forti perplessità per il metodo seguito. Sta alla maggioranza, Presidente, procedere con senso di responsabilità, evitando pasticci e confusioni. La nostra posizione è dunque legata all'atteggiamento della maggioranza e del Governo ed alla loro capacità di confrontarsi in quest'Aula, di non costringere il Senato ad un mero atto di ratifica ad ogni costo che rifiutiamo e respingiamo.

Cosa c'entra, poi, la caccia con le direttive e le normative europee, visto che l'Italia si è già adeguata, per la materia in oggetto, nella passata legislatura? Sicuramente, è un'operazione mediatica che assomiglia sempre più ad un ben orchestrato tentativo per raggiungere quegli obiettivi che più di venti *referendum* tra nazionali e regionali non sono riusciti a centrare; un piano che finora era stato impostato soprattutto su una cinica contabilità dei cosiddetti incidenti venatori, gonfiati fino all'inverosimile con l'aggiunta di infarti, cadute accidentali, incidenti di macchina e quanto altro si poteva aggiungere, il tutto con lo scopo evidente di creare presso la pubblica opinione e alcuni politici poco informati un clima di allarmismo del tutto privo di qualsiasi fondamento obiettivo. A completare questa ostinata e subdola strategia abolizionista è poi intervenuto un improvvido rapporto del WWF, nel quale il suo storico presidente Fulco Pratesi ricorda a tutti gli italiani l'improponibile e faziosa equazione «cacciatore uguale bracconiere», quando tutti noi qui presenti sappiamo che non è così, dimenticando però che Verdi ed ambientalisti sono orientati a fare parchi ed aree protette quasi con l'unico scopo di limitare l'attività venatoria e specularne poi sulle entrate, tant'è che lo stesso WWF, in una relazione di qualche tempo fa, dichiarava: «Oggi molte aree protette sembrano più agenzie di turismo, grandi *pro* *loco*, siti per fiere e mercati, più che luoghi deputati alla conservazione ed allo sviluppo sostenibile». Ma c'è qualcosa di più delle caciotte e dei salami, cari colleghi, se è vero - com'è vero - che il dottor Franco Tassi, onnipotente direttore (peraltro licenziato in tronco) del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) e lo stesso Fulco Pratesi, in qualità di Presidente, sono stati condannati dalla Corte dei conti a restituire, rispettivamente, 900.000 euro l'uno 88.000 euro l'altro. All'origine del severo provvedimento, come si può leggere su «Panorama» del 29 gennaio del 2004 e sulla rivista «Duemila» del 16 febbraio 2004, ci sono: finanziamento illegittimo a enti privati, spese di missione all'estero e in Italia, non accompagnate da un minimo di rendicontazione, utilizzo abusivo di carte di credito intestate all'ente, uso a go-go di automobili di lusso, appartamenti e beni vari. Insomma, a sentire i rilievi mossi dalla Corte dei conti, sembra che mentre il direttore spendeva e spandeva, il Presidente ometteva di effettuare i doverosi controlli: alla faccia della tutela del territorio, cari colleghi! Negli ultimi mesi, però, ad una simile campagna si è unita anche l'azione potente e apparentemente inarrestabile delle forze di maggioranza nelle quali, come è ben noto a tutti, la componente della sinistra radicale e dei Verdi, è portatrice, da anni, di una ferrea volontà antivenatoria. Di questa posizione così intransigente, purtroppo, non mancano esempi eloquenti che hanno finito per determinare un clima di assoluta e immotivata ostilità, senza che si riesca ad intravedere uno spiraglio per soluzioni condivise. Già nel mese di giugno del 2006 era apparso chiaro che la nuova maggioranza non aveva alcuna intenzione di porre rimedio alla rischiosa situazione che si era venuta a creare in merito alla gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Per tali istituti comunitari, infatti, si optava per convalidare la scelta, fatta da un Ministro Verde sul finire degli anni Novanta, che li equiparava impropriamente alle aree protette, ignorando, o fingendo di ignorare, che l'Europa non ha mai e poi mai dato indicazioni così rigidamente restrittive; anzi, ha sempre ritenuto che l'esercizio venatorio può rappresentare un ausilio insostituibile per una equilibrata gestione di tali aree. Sulla scia di questa interpretazione, palesemente viziata dalla visione ideologica e distorta di una parte del Governo, si è arrivati alla estemporanea e affrettata predisposizione di un decreto-legge agostano (il famoso decreto n. 251), che, oltre a non essere mai stato convertito, ha prodotto frutti a dir poco avvelenati. Infatti, questo provvedimento, preso senza la minima concertazione preventiva, ha suscitato la reazione di una gran parte dell'associazionismo venatorio, che ha dato vita alla imponente manifestazione, peraltro estremamente democratica, composta, civile e pacifica, del 1° settembre scorso. Quasi tutto l'autunno è così trascorso nell'onesto, ancorché tardivo tentativo da parte del ministro De Castro, di ricucire uno strappo imputabile solamente all'arroganza di chi riteneva (e continua a ritenere) che in materia ambientale e venatoria si possa e si debba dire solamente una raffica di no. Molti di questi - va detto con estrema chiarezza - sono assolutamente aprioristici e motivati da personalissime e opinabilissime interpretazioni ideologiche. A sgombrare però il campo da ogni equivoco e fraintendimento, è stato l'atteggiamento assunto dalla maggioranza in occasione della trionfale galoppata in sede di finanziaria. Infatti, con grande stupore, che per qualcuno, più o meno in buona fede, si è trasformata in una cocente delusione, nel maxiprovvedimento hanno trovato posto due emendamenti che si possono definire maldestri, a sostegno del dilettantismo e della supponenza di questo Governo. Il fatto è che il Ministro dichiaratamente anticaccia - lo voglio citare - Pecoraro Scanio, è riuscito a compiere un vero e proprio colpo di mano avocando al suo Dicastero il potere di controllo sull'Istituto nazionale per la fauna selvatica che, saggiamente, la legge n. 157 del 1992 aveva sottoposto alla vigilanza *super partes* della Presidenza del Consiglio. Il risultato di questo *blitz*, perfettamente riuscito, è che, d'ora in avanti, il controllore sarà, di fatto, sotto la diretta autorità del Dicastero controllato, con buona pace della logica, della suddivisione netta e trasparente dei compiti, dell'autorità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e perfino della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri. Ma siccome sembra che l'appetito di potere dell'onorevole ministro Pecoraro Scanio sia insaziabile, nella stessa finanziaria è stato inserito anche un altro punto, con il quale si stabilisce che sia proprio il Ministero dell'ambiente a fissare suoi personali criteri, cui le Regioni dovranno attenersi nell'adempimento delle direttive comunitarie. L'unico a non accorgersi dell'estrema gravità di questa vera e propria prova di forza messa in atto dal Ministro dell'ambiente, sembra essere stato il presidente del Consiglio, onorevole Prodi. Non così è stato, invece, per il ministro Paolo De Castro che, in una giustamente risentita lettera, si rivolge al Capo del Governo, sottolineando la gravita dei due commi della finanziaria. Riguardo al primo, il comma 471, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali chiede al presidente Romano Prodi di coordinare una riunione con il Presidente della Conferenza delle Regioni e i due Ministri interessati: lo stesso De Castro e Alfonso Pecoraro Scanio. II Ministro ricorda che finora l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), operando in sintonia con la Presidenza del Consiglio, i Ministri di agricoltura e ambiente e le Regioni, ha garantito con la sua competenza grande equilibrio tra la componente venatoria e quella ambientalista. Dice il Ministro: «Un'esigenza che non è venuta meno, e il ripristino di un ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio e la condivisione della responsabilità di vigilanza col Ministro che ha la delega per la caccia, eviterebbe che la decisione adottata venisse interpretata dal mondo venatorio come il venir meno di garanzie di equilibrio che il Governo intende viceversa continuare ad assicurare». Per quanto concerne il secondo comma, il 1226, il ministro De Castro esprime gravi preoccupazioni per le Regioni. Egli dice: «Le Regioni non vengono in questo modo ascoltate e cade il concorso precedentemente previsto del Ministero delle politiche agricole Cari colleghi, considerato il clima sicuramente non pacifico, né tollerante, che si sta creando e alimentando sulla caccia, e che questi ultimi irrituali avvenimenti politici hanno messo ancor più in risalto, credo sia opportuno fare un minimo di chiarezza su una problematica così complessa che solo una visione radicale ritiene di poter ricondurre allo stantio dilemma: caccia sì, caccia no. Ovviamente, nessuno ignora che i cacciatori rappresentino una minoranza nella moderna società. Ma questa minoranza è pur sempre costituita da 800.000 iscritti, (dobbiamo calcolare anche il loro indotto familiare), onesti, anzi, integerrimi cittadini, che hanno gli stessi doveri e che dovrebbero avere gli stessi diritti di tutti gli altri. però non sembra essere. Tanto che gli appassionati dell'arte venatoria avvertono un totale disinteresse e una crescente indifferenza politica nei loro confronti. Vediamo di non creare anche il Partito dei cacciatori all'interno di questo Parlamento. E tutta questa ostilità, che, come ho già sottolineato, è più preconcetta che solidamente e scientificamente motivata, sta raggiungendo il suo culmine proprio in un momento in cui i cacciatori hanno preso, di sé e della loro attività, una coscienza diversa e sicuramente più moderna. fino al punto da trasformarsi in veri e propri gestori e tutori dell'ambiente, oltre che in guardiani attenti e motivati del comune patrimonio naturale. Basti pensare al grande lavoro svolto in collaborazione con Protezione civile e Corpo forestale dello Stato, per il tempestivo avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi; o la totale disponibilità offerta alle autorità competenti per monitorare quotidianamente ogni più sperduto angolo di territorio; ricordo il lavoro che è stato fatto dai cacciatori quando c'è stata l'emergenza dell'influenza aviaria. Addirittura il recupero di sentieri, delle pozze d'abbeverata, lo sfalcio dei terreni montani non più pascolati. Proprio per questo, ritengo sia doveroso richiamare l'attenzione di tutti i colleghi verso un così gran numero di cittadini e sulle loro esigenze, rese peraltro pienamente legittime dalla vigente normativa internazionale e dalla quasi totalità degli scienziati e dei tecnici che si occupano di protezione e gestione della fauna selvatica. In ballo, però, non ci sono solamente il rispetto per la dignità altrui, o la sacrosanta difesa di tradizioni millenarie e di una sana cultura rurale. Accanto a questi aspetti puramente culturali e antropologici, coesistono anche i valori economici, occupazionali e sociali di un gran numero di di un gran numero di lavoratori che operano sia nella produzione di armi e munizioni sportive, sia in un indotto quanto mai vasto, che spazia dalla buffetteria al turismo, dalla veterinaria all'oggettistica: in particolare è da rilevare che l'impatto economico totale è di euro 2.150 milioni e che gli addetti dell'intero settore, comprensivi dell'indotto, ammontano a circa 50.000 unità. Cari colleghi, ci sembrano cifre sulle quali tutti, associazioni venatorie, ambientalisti, politici, *mass* *media* e opinione pubblica dovrebbero meditare. Ritengo che tutti Ritengo che tutti noi che siamo stati chiamati dalla volontà popolare a gestire la cosa pubblica, dobbiamo sentire l'obbligo morale di considerare, con la massima attenzione, le legittime istanze di milioni di cittadini, isolando ogni forma di intolleranza e ricercando, con coerenza e onestà intellettuale, civile e sociale, quegli stessi compromessi che non solo stanno rendendo possibile la sopravvivenza della caccia in tutte le più moderne società, ma anzi l'hanno elevata ad attività indispensabile per una corretta gestione ambientale. *(Applausi

- che è uno dei punti contenuti nel provvedimento che stiamo esaminando - siamo nelle condizioni di porre il nostro sistema bancario al passo con la concorrenza europea ed internazionale, ma anche di rendere finalmente più trasparenti le modalità di relazione che intercorrono tra il sistema bancario e il tessuto delle imprese. Il sistema di valutazione, basato su un *rating* interno trasparente, potrebbe permetterci di superare due dei limiti maggiori del nostro sistema bancario: da un lato la grande difficoltà per il tessuto di piccole e medie imprese, che formano l'infrastruttura economica del Paese, nell'accedere al credito bancario; dall'altro, la mancanza di trasparenza nella sottoscrizione di investimenti da parte dei piccoli investitori, delle famiglie e dei lavoratori. Per quanto riguarda il primo aspetto (l'accesso al credito), siamo di fronte ad una vera e propria urgenza: la sottocapitalizzazione del nostro sistema produttivo è un dato noto che però, di fronte alla sfida del mercato globale, diviene un grande limite. È convinzione diffusa che le leve per la crescita siano ricerca ed innovazione e ciò richiede ingenti investimenti; ma solo attraverso questo impegno da parte delle imprese sarà possibile competere con la qualità al vero e proprio *dumping* sociale fatto da alcuni Paesi che preferiscono scegliere la diminuzione del costo del lavoro e la negazione dei diritti dei lavoratori. Ciò che deve essere chiaro è che l'Accordo Basilea 2 non può diventare un alibi per togliere al sistema bancario le proprie responsabilità. La scelta di dare credito a vere e proprie rendite finanziarie, come è accaduto negli ultimi anni nel mercato immobiliare a scapito del sistema produttivo, non può essere giustificata attraverso il riferimento a quell'Accordo. Per quanto riguarda il secondo aspetto, non credo sia necessario ricordare in questa sede vicende come Parmalat o i *bond* argentini, vicende in cui i piccoli risparmiatori hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita. Il rafforzamento del ruolo della Banca d'Italia e delle procedure di coordinamento tra le varie strutture europee, può essere un freno a tale modello, che fa dei piccoli risparmiatori piccoli risparmiatori carne da cannone nel gioco della finanza. Anche qui, però, alle norme devono conseguire i comportamenti delle autorità preposte al controllo, che ora vediamo affidate in mani più sicure delle precedenti.

su un decreto che contiene provvedimenti tra loro eterogenei. Tuttavia, se andiamo a fare una valutazione di merito sui singoli interventi, vedremo non solo come i criteri di necessità ed urgenza vengano pienamente soddisfatti, ma vedremo, soprattutto, come la positività di queste scelte faccia venir meno ogni perplessità. Le norme contenute negli articoli 4 e 5, infatti, rispondono a vere e a proprie emergenze. L'articolo 4, sospendendo le deroghe previste dalla Regione Liguria sulle tipologie di specie animali che possono essere cacciate, consente di limitare un danno che sarebbe stato incalcolabile rispetto ad alcune specie a rischio di estinzione. Si definisce, quindi, confermato dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per il quale non possiamo ammettere deroghe indiscriminate, se non vogliamo mettere in discussione la biodiversità presente nel nostro Continente. La crescita incontrollata delle aree di antropizzazione ha già creato abbastanza danni e siamo convinti che non sia utile consentire ad una attività ludica, quale la caccia, di mettere ulteriormente in difficoltà l'ambiente in cui tutti noi viviamo. Un altro aspetto che deve essere valorizzato è l'istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani, che non solo sostituisce la precedente Agenzia nazionale italiana gioventù, ma comincia ad assumere una maggiore autonomia dalla precedente. precedente. Dopo l'approvazione del provvedimento che stiamo discutendo, speriamo di non assistere semplicemente ad un aggiustamento burocratico delle competenze tra i Ministeri, ma ad un vero e proprio rilancio di questo fondamentale strumento. L'Agenzia, infatti, ha due compiti prioritari: la gestione del programma comunitario Gioventù in azione e il supporto alle attività del *Forum* dei giovani. Quando fu istituito, nel 2004 il *Forum* dei giovani è stato uno degli ultimi organi di questo tipo approvati tra i diversi Paesi della Comunità Europea. Ma ancora questo luogo non riesce a dare il segno vero delle domande e delle aspettative dei giovani del nostro Paese. Tutto ci serve tranne che una piccola palestra politica che tenti di riprodurre le Aule parlamentari. Serve invece un luogo che sappia dare il segno delle domande di questo pezzo di società: penso ad esempio all'enorme tema dell'autonomia abitativa dei giovani. Come noto, nel nostro Paese il 70 per cento dei giovani fino a 35 anni vive ancora in famiglia. E questo non avviene certo perché i ragazzi italiani siano, come si dice, mammoni: avviene per precise ragioni economiche legate da un lato lato alla precarizzazione dei rapporti di lavoro e dall'altro ad un mercato immobiliare che non reputa più la casa un diritto, ma solo una rendita. Quel *Forum* dovrebbe costituire un monito per tutte le istituzioni affinché pongano al centro queste fondamentali dovrebbe essere il luogo istituzionale che indica la strada per costruire il futuro delle giovani generazioni. Questo, purtroppo, fino ad ora non è avvenuto. L'altro aspetto rispetto al quale ci aspettiamo molto dall'Agenzia è quello del ruolo dell'Italia nel programma Gioventù in azione: è attraverso strumenti come questo, o come il più noto «Erasmus» che si costruisce l'idea di una cittadinanza europea, necessità oggi sempre più urgente di fronte ai limiti di una politica che intende l'Europa non come identità e comunità, ma solo come mercato. Gli anticorpi ad una deriva mercantile dell'idea di Europa stanno proprio in questi ragazzi che, sacco a pelo in spalla, girano per questo nostro grande continente Sono questi alcuni motivi di merito che ci consentono di valutare positivamente un provvedimento di certo eterogeneo, ma necessario ed urgente non solo per rafforzare il nostro tessuto produttivo, ma anche per dare nuove prospettive alle giovani generazioni

l'Italia e il recepimento di Basilea 2; le eccezioni mosse a livello internazionale; i rapporti tra Governo e opposizione. Come sappiamo, l'Italia è tra i Paesi che, dalla fine dell'anno passato, rispettato i termini di recepimento della direttiva sui requisiti patrimoniali. Tale direttiva comprende al suo interno l'Accordo di Basilea, che che si fonda su principi di duttilità e trasparenza. È chiaro che il nuovo assetto che si va delineando è fondato sulla stabilità delle banche e dunque del sistema bancario nel suo insieme: sul «come», cioè, sia possibile valutare e calcolare adeguatamente il coefficiente di rischio rispetto alla trasparenza dei bilanci delle aziende che usufruiscono del credito. Sarà bene notare che nella trasposizione italiana della normativa, guardando ad istituti di credito di media o considerevole grandezza, si è tenuto conto della specificità del nostro sistema bancario, con particolare riferimento alla fascia medio-piccola. In che modo? Considerando i parametri essenziali a tal fine, quali l'adeguatezza patrimoniale (maggiormente garantita da una previsione e da una programmazione pluriennale) o i fattori macroeconomici avversi (di cui sono stati analizzati i possibili impatti). L'Accordo di Basilea rappresenta, dunque, uno snodo essenziale per il rapporto tra banche e imprese e dunque per lo sviluppo. Non solo si è cercato di lavorare nel solco di una maggiore equità, agendo sulle differenziazioni tipologiche interne al sistema, ma si è fornito nuovo alimento a quei settori di sviluppo in cui più fortemente si avverte il ruolo della ricerca e della sperimentazione di soluzioni innovative, intervenendo sulla quantificazione dei rischi e sull'adeguatezza patrimoniale nella sua valutazione prospettica. È chiaro che le banche - per far fronte nel migliore dei modi alla necessità di adeguarsi alla normativa - già da tempo hanno aperto un'approfondita riflessione sulle modalità del cambiamento, ma sarebbe una scelta miope attardarsi e non affrontare quelli che appaiono sempre più, in un quadro macroeconomico fluido, attraversato da incertezze, fattori competitivi determinanti quali una più attenta e raffinata capacità di gestione dei rischi e le scelte in termini di governo aziendale che ne derivano. La disciplina dell'Accordo di Basilea ha indicato una serie di linee guida cui adeguarsi, ma senza per questo cadere nel ristagno e nelle ischemie che talvolta costituiscono il criterio ispiratore del dettato e che vi sottostanno. In altri termini, a un'assenza di eccessiva prescrittività si è coniugata una sostanziale capacità volta a sapersi muoversi, senza stravolgere, su quelle che possono essere considerate linee guida accettabili e prassi ritenute ormai in uso dagli intermediari, favorendo fra l'altro una maggiore trasparenza. Un punto fondamentale è che il nuovo Accordo di Basilea ha come fine quello di armonizzare la normativa su scala globale: vale a dire che i parametri non mutano a livello internazionale e sono validi quindi per tutto il mondo, eccezion fatta dagli Stati uniti d'America, che si sono opposti al provvedimento per quel che concerne le piccole banche. Certo, è da considerare la specificità del sistema bancario statunitense, ispirato da criteri di maggior liberismo; tuttavia destano perplessità simili posizioni e resistenze. Mario Soldati scriveva che fra tutte le forme di lontananza l'America rimane la più vera e autentica. Non sono certo antiamericano, appartengo a una generazione che si è specchiata nella cultura e nei miti americani (dal cinema, alla musica, alla letteratura e anche alla politica), ma che ora fa sempre più fatica a rispecchiarvisi. Non si è nel torto, a mio avviso, nello stigmatizzare un ormai proverbiale «*Yankee go home*», troppo spesso affrettato; tuttavia, l'America ci ritorna, fuori dai brillanti riti, anche attraverso il rifiuto di aderire al Protocollo di Kyoto (i cui danni sono incalcolabili, anche per le derive morali verso India e Cina), la strage del Cermis (il pilota - come ricordiamo - fece ritorno in patria, ottenendo una promozione dopo pochi mesi) e, da ultimo, il *marine* Lozano (imboscato fra le ballerine di fila in una base imprecisata e senza possibilità di estradizione). Spiace dover ammettere che non è un bello spettacolo, anche se osservato dall'estrema periferia, da un'Italia che assomiglia sempre più alla brutta copia di una brutta America, di un'America che spesso è concentrata su sé stessa e che appare in molti casi lungi dal comportarsi come la grande nazione che merita di essere valutata. Uno fra gli obiettivi fondamentali dell'Accordo di Basilea 2 è l'obbligo, da parte degli intermediari e delle banche, a informare il mercato sui parametri di rischio e adeguatezza patrimoniale, in modo tale che anche la clientela possa indirizzarsi verso le banche più efficienti. Tanto più le eccezioni sollevate dal centro-destra in Commissione mi paiono strumentali e sostanzialmente prive di fondamento: una conferma, se ce ne fosse bisogno, di un'opposizione che troppo spesso sa guardare soprattutto alla convenienza dei numeri e solo in parte al bene del Paese. Faccio notare, a tal proposito, che alcuni emendamenti riguardanti l'Agenzia nazionale per i giovani - ne hanno parlato alcuni colleghi - bocciati in Commissione, sollevano una questione reale, com'è quella dell'inserimento delle nuove generazioni (in particolare delle donne) nel mondo del lavoro. Credo che il relatore, senatore D'Amico, abbia già predisposto un ordine del giorno nel quale vengono riassunte le proposte avanzate a tal fine.

dove l'opposizione non ha determinato condizioni per porre in essere una politica strumentale (correggo sotto tale aspetto il collega che mi ha preceduto). L'opposizione è stata invece costretta ad abbandonare l'Aula a causa di due ragioni e di due motivi fondamentali: l'importanza del problema, che avrebbe imposto tempi sicuramente più ampi di discussione e di analisi, e la chiusura a riccio premeditata, preordinata, aprioristica, da parte della maggioranza a qualsiasi modifica, sia pure di tenore migliorativo. Il testo giunto al Senato sotto forma di decreto‑legge non solamente è privo delle caratteristiche di urgenza, ma anche di omogeneità tra le varie materie presenti nel provvedimento: prelievo venatorio, Agenzia nazionale per i giovani, assistenza a terra negli aeroporti.

penserebbe di trovarsi di fronte a soggetti che recitano ognuno una parte diversa. C'è chi discute dell'Agenzia per i giovani (ritornerò su questo punto), c'è chi discute dell'ipotesi dell'assistenza a terra negli aeroporti, c'è

tuttavia ricordare a chi è presente in quest'Aula, ma soprattutto a chi probabilmente è affascinato da una certa teoria dell'occupazione (o meglio della disoccupazione), che la realtà a cui ha fatto riferimento poco fa non è più quella.

di far imboccare a tutti loro la strada giusta verso l'occupazione e l'inserimento sociale. Ma ti sfugge un fatto: ci sono oggi, in questa nostra Italia, fasce e e segmenti di quarantenni e di cinquantenni che non riescono a trovare un posto di lavoro e che soprattutto, non essendo in possesso (non per colpa propria) di un'adeguata qualificazione, non avranno mai alcuna prospettiva di lavoro. Ebbene, non una parola è stata spesa in questa direzione, nonostante si tratti normalmente, a differenza dei cosiddetti giovanissimi, di soggetti, di gente, di cittadini, di potenziali lavoratori che hanno alle spalle nuclei familiari, senza sapere quale potrà essere il futuro non solamente del capo famiglia, ma del nucleo familiare medesimo. Sarebbe stato pertanto opportuno trattare monotematicamente tutti questi problemi, creando le condizioni e i presupposti per un'analisi seria, puntuale, capace di indicare obiettivi ben precisi.

avrebbe imposto una riflessione sulla natura giuridica delle direttive medesime. Queste non sono equiparabili ai regolamenti. I regolamenti hanno la funzione di rendere omogenei gli ordinamenti giuridici per le parti interessate e quindi di creare le condizioni di un sostanziale diritto comune; le direttive hanno un'impostazione e una natura giuridica diverse, quelle di avvicinare, sia pur gradualmente, situazioni differenti tra Paese e Paese, creando le condizioni per tener conto necessariamente delle specificità. Quando parleremo delle piccole e medie imprese in riferimento a Basilea 2, cercherò di dimostrare che la situazione delle piccole e medie imprese nel nostro Paese, nella nostra Italia, è completamente diversa da quella esistente in altri Paesi europei. Che bisogno c'era dunque di procedere a tappe forzate? Che bisogno c'era di evitare una riflessione collegiale, visto che, almeno su questo tema, ne va della situazione socio‑economica del Paese, ne va - io dico - dell'intero sistema Paese? Vorrei ricordare qualcosa di Basilea 2, partendo, sia pure rapidamente, da Basilea 1. Gli Accordi di Basilea 1, risalenti al 1998, prevedevano sostanzialmente un sistema di garanzie standardizzato, in virtù del quale gli istituti di credito concedenti prestiti erano obbligati ad accantonare una percentuale fissa delle somme prestate sulla base della natura delle categorie richiedenti, divise fra quelli a maggiore o a minor rischio. Tutto questo senza che vi fosse riferimento alcuno all'effettiva solvibilità della controparte. Era un passaggio, si costituiva un fondo, però non si arrivava alla definizione complessiva del sistema al quale saremmo e siamo giunti con Basilea 2. con il nuovo accordo sancito dal comitato di Basilea, organismo del quale fanno parte i rappresentanti delle Banche centrali dei maggiori Paesi, sono state stabilite regole nuove e molto più rigorose sui requisiti patrimoniali delle banche, sintetizzabili nei cosiddetti tre pilastri, cioè il nuovo metodo di calcolo del rischio del credito, le modifiche della supervisione degli organi di vigilanza delle Banche centrali, il ricorso alla disciplina del mercato mediante la trasparenza informativa. Qualcuno probabilmente avrà pensato che questa normativa di Basilea 2 tocchi e interessi esclusivamente le banche, ma non è così: parte interessando inizialmente le banche, ma poi si trasferisce a macchia d'olio sull'intero sistema socio‑economico del Paese. Questo Questo accordo entra in vigore nel 2007, ma ho evidenziato poco fa la differenza fra i regolamenti e le direttive. Avremmo avuto la necessità di creare le condizioni che su Basilea 2 si determinassero

non solamente un pezzo importantissimo dell'economia, ma anche decine o forse centinaia di migliaia di posti di lavoro. ora gli effetti di Basilea 2 sull'impresa. Se è vero che Basilea 2 incide prevalentemente sul sistema organizzativo e decisionale delle banche, costringendole a quantificare e supportare ogni attività bancaria con una sorta di capitale di vigilanza, capace di coprire e garantire l'assunzione di un certo grado di rischio, è altrettanto vero che tali disposizioni esplicano i propri effetti anche, o forse soprattutto, sull'impresa, su tutte le imprese in via generale, al di là delle dimensioni delle stesse, ma in maniera più pesante sulle piccole e medie.

non solamente la vita passata e presente, che serve per l'analisi, ma anche quella futura dell'azienda, che serve per la sintesi. Una trasparenza non rigida, ingessata ma dinamica, capace cioè di affrontare l'analisi dei bilanci, l'andamento dei crediti e dei debiti, l'eventuale criticità del rapporto bancario, ma anche

(una sorta di riassicurazione, come i manuali di diritto commerciale insegnano), fattori indispensabili nella valutazione del rischio. Sicché automaticamente verrebbe a determinarsi una sorta di selezione tra le imprese virtuose e meritevoli, che quindi godranno di condizioni molto favorevoli all'accesso al credito, e quelle meno solide e trasparenti, che, da un lato, vedranno crescere l'onerosità della loro esposizione e, dall'altro, potrebbero trovarsi completamente fuori mercato. con Basilea 2 la valutazione della rischiosità dell'affidamento bancario, al di là del fatto che potrà essere indirizzato, tenuto, portato avanti o gestito da importanti agenzie specializzate per il *rating* esterno, potrà contare anche sul cosiddetto *rating* interno. Ma, in qualsiasi caso, il rischio rimane e oggi vorrei chiedere ai colleghi della maggioranza se si sono posti qualche problema. Infatti, nonostante alcuni istituti di ricerca e la stessa Commissione europea si siano espressi ottimisticamente sulle dinamiche

richiesti alle banche rispetto agli attuali, quindi una sorta di sostanziale arretramento, non c'è dubbio che le piccole e medie imprese, operanti soprattutto (lo dico sottovoce) nell'Italia meridionale, dovranno fronteggiare non poche difficoltà. sottocapitalizzazione: è vero o non è vero che la maggioranza delle piccole e medie imprese meridionali è sottocapitalizzata? Si risponda sinceramente, serenamente, lealmente, a questa domanda. difficoltà di costanza e di coerenza della redditività aziendale: quante sono le imprese che chiudono con il conto economico in situazione positiva?

un'impresa sottocapitalizzata e priva di redditività non può determinare le condizioni per poter modificare se stessa in maniera strutturale. E allora, se ci sono queste fragilità che, a mio avviso, appaiono insormontabili,

si sarebbe dovuto fare. Il Governo doveva venire qui a dire: o assistiamo passivamente alla demolizione di questo sistema d'impresa oppure creiamo le condizioni per poter sostenere adeguatamente il passaggio da una fase in cui la discrezionalità delle banche e degli intermediari finanziari era massima e molto dipendeva dalla valutazione (molto soggettiva) del rischio che poteva fare il gestore, il titolare, del potere decisionale all'interno dell'istituto di credito, ad una fase nuova, in cui si passa ad un regime quasi ragionieristico o da scienza esatta. Si sarebbe dovuto fare altro. Ai signori del Governo vorrei chiedere: avete pensato a tutto questo, è stato fatto qualcosa? Avete creato le condizioni per sostenere con risorse adeguate, per esempio, la fornitura di servizi reali miranti alla modernizzazione strutturale dell'impresa senza che tutto ciò incidesse sull'indebitamento?

del sistema economico italiano in generale e meridionale in particolare vi è anche la farraginosità del sistema burocratico alla quale bisogna dare sicuramente una risposta in tempi brevi?

si troveranno fuori mercato, non avranno più la possibilità di intervenire strutturalmente sul territorio. Altro che occupazione: saranno costrette sostanzialmente a chiudere. E allora, una volta tanto, a voi che avete accusato il centro-destra di essere affezionato alle sanatorie,

dei bisogni e delle specificità del territorio; un provvedimento che sostanzialmente è il frutto della vostra incapacità politica, allora, fatela, fatela subito, perché anche nei prossimi giorni noi batteremo molto su questo tema creando le condizioni per sensibilizzare il sistema economico sui rischi che sicuramente si corrono. in questo momento governate, al vostro Governo, su cui ricade la più grande responsabilità politica dei drammi che potrebbero venire a determinarsi nel prossimo futuro, la responsabilità delle prossime ore, quando discuteremo degli emendamenti, prima delle dichiarazioni di voto, prima del licenziamento del provvedimento, di poter chiudere in maniera un po' più gloriosa

Presidente, colleghi, mi viene in mente un'espressione di un mio maestro in politica, quando all'orizzonte compariva la fragilità delle economie e delle politiche degli Stati europei e

Egli concludeva un suo comizio dicendo «Dobbiamo pensare alla riforma delle riforme, ovvero a realizzare l'Unione Europea»: per onore di autore, l'espressione era del professor Giuseppe Codacci Pisanelli. Egli, già a quell'epoca, come la classe politica di allora, aveva capito che agganciare l'Italia all'Europa era la soluzione ideale per un Paese come il nostro, che mostrava limiti sul piano organizzativo, strutturale, economico e sociale. La "riforma delle riforme" sembra oggi quasi un'espressione da vate

Allora, siamo consapevoli dell'anemia del sistema produttivo italiano, peraltro più accentuata di quella di altri Paesi - si pensi alla Germania

sul risultato economico delle aziende in misura sensibilmente più lesiva in Italia di quanto non accada negli altri Paesi, dove il tasso di indebitamento medio del sistema è molto più basso. E allora, siamo consapevoli che a noi è dato un compito più arduo,

il sistema bancario del Mezzogiorno non avrebbe mostrato limiti e non si sarebbe verificata la sciagurata soluzione della settentrionalizzazione, nel malinteso di evitare gli scandali e non considerando colpevole il sistema bancario, ma erano le tossine del sistema produttivo scaricate sul sistema bancario che un Governo oltremodo interessato e interessante avrebbe dovuto rimuovere, per non togliere

pur con la loro virulenza, alla quale ha fatto riferimento il senatore Curto, non avremmo avuto questa grande sciagura. Allora, ben venga la riforma delle riforme alla quale faceva riferimento il mio maestro; ben venga l'applicazione di queste norme, ma sia chiaro: verrà una nuova stagione; le stagioni si avvicendano. Non ci sarà sempre un Governo, che non riesce a parlare al suo interno; non ci sarà un Governo che non può prestare attenzione a quello che accade tutto intorno; verrà certamente un Governo che saprà tenere conto delle difficoltà del sistema produttivo in costanza di applicazione di queste rigorosissime norme che si riveleranno in principio come una sorta di ingessatura del sistema produttivo e non potrà andare oltre i limiti, perché il sistema bancario necessariamente dovrà fare i conti con i propri rendiconti e dovrà tenere conto anche di un minimo di flessibilità da praticare. ed è possibile praticare la flessibilità per poter consentire che questo nostro sistema produttivo si adegui a queste esigenze di rigore, che io ritengo necessarie ed indispensabili per evitare che ulteriori sciagure si abbattano questa volta non soltanto sul sistema produttivo meridionale, ma su quello nazionale. Allora, ben venga la riforma delle riforme ed il Governo sia grato ai padri che postularono l'esigenza di realizzare l'integrazione europea perché senza queste norme oggi, quest'Italia, che non ha Governo, che ha un Governo che non riesce a parlare nemmeno con se stesso, come avrebbe fatto?

delle direttive comunitarie, note Basilea 1 e Basilea 2, che costituiscono l'asse portante del decreto-legge varato il 27 dicembre, in tempo utile rispetto alla scadenza del 31 dicembre; decreto-legge che ha consentito immediatamente alla Banca d'Italia di renderlo applicativo con una sua circolare. questo decreto-legge un atto dovuto: era atteso dal mercato, era atteso dagli operatori economici. Di cosa si tratta in particolare? Di omogeneizzare le regole di vigilanza, prudenziale sulla stabilità degli intermediari; di definire dei criteri omogenei per evitare forme di concorrenza nociva, sleale, per definire degli *standard* minimi uniformi. Insomma, nel quadro delle iniziative che costruiamo in Europa - perché io penso che dobbiamo valorizzare questo aspetto che ci deriva da questa Comunità nella quale operiamo fare in modo che il mercato, la sua crescita si coniughino con la trasparenza e la informazione al pubblico. È avvenuto così, con l'attuazione della *market abuse*; deve avvenire così, superando il pasticcio con l'attuazione della MiFID, con l'attuazione della direttiva sull'OPA. Insomma, abbiamo la necessità che si rendano più precisi i metodi per misurare i rischi assunti dalle banche. Occorre, cioè, definire un parametro ragionevole per valutare l'adeguatezza patrimoniale in relazione ai capitali vincolati. Tutti ricordiamo le preoccupazioni, i dubbi, le sofferenze all'epoca di Basilea 1. Ora Basilea 2 migliora le procedure di valutazione del rischio del credito in una misura - e poi ci tornerò - che è più favorevole per il sistema delle piccole imprese. Tre sono i criteri, le novità che sono meglio articolate e meglio definite. Il rischio non è più valutato per classi di strumenti finanziari, ma è proporzionato il vincolo di capitale a rischio assunto rispetto al singolo cliente. Ancora, le società di *rating* possono essere utilizzate dagli intermediari finanziari, che possono anche acquisire informazioni sui rischi, utilizzando delle metodologie che devono essere delegate dalle autorità di vigilanza. luogo, la valutazione è riferita oltre ai rischi, anche al cambio e agli interessi. Pertanto, l'attuazione di tale direttiva viene incontro alle piccole imprese. Abbiamo una particolare sensibilità nei confronti delle piccole imprese; non facciamo della propaganda. Nella legge finanziaria, nella strategia generale del Governo della maggioranza, diamo molta importanza alle piccole imprese, perché sappiamo che esse sono una parte essenziale della ripresa che si sta consolidando nel Paese e che vogliamo rendere strutturale, perché sappiamo che attraverso le piccole imprese, il sostegno alla loro competitività, diamo anche una risposta importante ai problemi dell'occupazione e della buona occupazione. Ecco perché tali misure si inquadrano nelle altre che abbiamo preso: mi riferisco alla soluzione che è stata trovata sul trattamento di fine rapporto, che non è optato; mi riferisco

infatti, che la scommessa per il futuro del nostro Paese è di sostenere la straordinaria particolarità rappresentata da questo mondo. Abbiamo anche migliorato il sistema dei cofidi. Sappiamo che non tutto è risolto, che bisogna arricchire lo spettro degli interventi che devono essere adottati a questo riguardo e che si possono esplorare altri strumenti, sapendo qual è il problema delle piccole imprese, la possibilità delle cambiali finanziarie, la possibilità di emettere obbligazioni, la possibilità di esplorare anche un sistema di borse locali. Venendo al problema delle piccole imprese, di Basilea 2 e di questa direttiva comunitaria, il relatore, il senatore D'Amico, con grande competenza ed efficacia ha smentito quel luogo comune che abbiamo sentito ripetere ancora nel dibattito. Abbiamo sentito parlare di elefanti che entrano nei negozi di cristalleria;

e minori capitali da accantonare per la copertura dei prestito richiesti, perché a parità di volumi di crediti erogati si tiene conto del numero e della qualità dei soggetti finanziati.

soltanto tecnico: si tratta di un provvedimento di grande impatto economico, perché sostiene la ripresa e si inquadra in una strategia dove la tecnica è messa dalla politica al servizio dello sviluppo.

la ristrettezza dei tempi è stata tiranna e non abbiamo potuto fare questo confronto. Queste preoccupazioni, però, queste considerazioni che ha fatto l'opposizione e che erano presenti anche negli interventi di alcuni di alcuni colleghi, in particolare del senatore Barbolini, vanno considerate. Mi rivolgo al sottosegretario Tononi noi abbiamo bisogno di ricercare il confronto: non bisogna evitare il confronto in Aula, è fondamentale che il Governo organizzi i tempi e le procedure, di modo che in Parlamento - e io parlo qui al Senato

gli rivolgo la raccomandazione di farsi interprete con il Governo di queste istanze. Abbiamo da rimediare il pasticcio della MiFID, abbiamo la direttiva sull'OPA, c'è bisogno che si discuta, che ci sia questo confronto anche con l'opposizione.